vengono elencati i nomi dei senatori che intervengono sul punto, che - se ben ricordo - sono i senatori Calderoli, Boccia, Castelli, Schifani

La ringraziamo, senatore Malan, le sue osservazioni sono assolutamente pertinenti, dovendosi trattare degli atti, delle deliberazioni, dell'oggetto della discussione e di chi vi ha partecipato. Il processo verbale verrà quindi

è avvenuto per la costituzionalità dell'atto Senato n. 741, il cosiddetto decreto-legge Visco-Bersani, si sta ripetendo per altri provvedimenti,

e che invece non sono stati utilizzati, nonostante la richiesta dell'opposizione. Signor Presidente, dico questo perché in particolare

non ha potuto tener conto delle osservazioni della 1a Commissione. Ora, Presidente, capisco l'ingolfamento dei lavori, il periodo prefestivo, eccetera, però credo che licenziare un Documento come questo senza un'indagine approfondita in Commissione relativamente ai due settori strategici della manovra che il Governo intende basare poi sul Documento di programmazione economica, di programmazione economica, sia estremamente grave. Voglio aggiungere, Presidente, e di questo mi sono reso conto proprio recandomi questa mattina di buon'ora in 5aCommissione per far presente l'assenza di tale parere,

non abbiamo avuto l'opportunità di partecipare nemmeno in discussione generale alla formazione dei convincimenti della maggioranza, che avrebbe dovuto ma non ha

con l'Ufficio di Presidenza senza che particolari richieste siano state avanzate, se non quelle poi inserite all'ordine del giorno.

la discussione sui vari punti è stata incardinata, si è svolta, e, poi, dal momento in cui sono ripresi i lavori d'Aula, non si è potuto procedere al voto. Infine, per quanto riguarda il parere sul DPEF, quel documento di cui il senatore Pastore è entrato in possesso non è affatto un parere, perché non è mai stato approvato dalla Commissione. Immagino si tratti della bozza di parere

per così dire, ufficiale, non era dimenticato su un banco. BALDASSARRI *(AN)*. Era a fianco di altri documenti. Anche noi, come Commissione bilancio, ieri non abbiamo potuto completare i lavori, data la concomitanza dei lavori in Aula. Faccio però presente al presidente Bianco che il presidente Morando ha convocato la Commissione bilancio questa mattina alle ore 7 proprio per essere in grado di completare i lavori entro le ore 9,30 per l'apertura della seduta in Aula. Questo non impediva alle altre Commissioni di fare Sull'ordine dei lavori, invece, signor Presidente, ho chiesto in chiusura di seduta della 5ª Commissione al presidente Morando, che mi ha dato una precisa risposta, se è disponibile è disponibile per le Commissioni, ma soprattutto per l'Aula, da parte del Governo, la tavola relativa al conto economico delle pubbliche amministrazioni-andamento programmatico. A questo momento esiste solo la tavola con l'andamento tendenziale a legislazione vigente. Ricordo che si tratta di una prescrizione di legge e che il DPEF non può essere considerato completo senza la documentazione riferita a questa tavola. Al di là della formalità normativa, c'è poi il fatto che l'andamento programmatico della finanza pubblica da qui al 2011 è il cuore portante del DPEF. Questa tavola, al momento, è indisponibile è indisponibile per la Commissione e per l'Aula. Non so se questa può essere una pregiudiziale, però certamente il Governo è tenuto a presentarla in Aula.

ho qui il calendario indicativo dei lavori della Commissione - per la giornata di ieri il DPEF non era previsto: la posizione della questione di fiducia e la conseguente sconvocazione delle Commissioni non hanno influenzato l'andamento della discussione sul DPEF che, a mio ricordo, si è invece fermata alla sola esposizione da parte del relatore.

il rapporto con il tendenziale e gli obbiettivi programmatici, quindi da questo punto di vista la richiesta del senatore Baldassarri è stata già esaudita in sede di predisposizione del DPEF. Il senatore Baldassarri si preoccupa della mancanza nel DPEF del conto delle pubbliche amministrazioni programmatico, che effettivamente è cosa parzialmente diversa dalla tabella cui ho fatto prima riferimento.

ha fatto riferimento. Dire che negli anni passati non è stata mai presentata significa affermare che c'è stato un mancato rispetto della legge nel passato, che continua anche in questo momento.

*(Ulivo)*. Signor Presidente, credo che tutto sia stato chiarito. Però, se è vero che ci sono questi precedenti e se è vero, come giustamente il senatore Morando ha fatto rilevare, che comunque nel DPEF ci sono i dati, vorrei riconoscere che il collega Baldassarri non ha tutti i torti. In passato, in presenza di richieste

posto questioni pregiudiziali di procedura, quindi con molto senso di responsabilità. Voglio dargli atto di questo e chiedere cortesemente

forma, ma la sostanza. Quindi, una tabellina, nel corso della giornata, prima che si proceda al voto sul DPEF: se il Governo fosse in grado di fornire

Mi rendo conto delle difficoltà, ma credo che il Governo sia in grado con i suoi uffici, nel corso della giornata, prima del voto, di fornire quel minimo quadro di riferimento, quell'informazione, quell'informazione, che oggettivamente rende il voto più trasparente. Non credo di chiedere al Governo, unitamente al collega Baldassarri che ha avuto questa esperienza e che sa che si può fare,

esprimere la mia opinione su alcune questioni che sono emerse. Stiamo vivendo giornate un po' concitate

che hanno ripreso una vecchia polemica: il DPEF non serve a niente, stiamo facendo, in fondo, un esercizio verbale, retorico; la maggioranza, il Governo, il Parlamento, decideranno di cancellare questa parte di procedura nella formazione del bilancio e della manovra di finanza pubblica, meglio sarà. Un autorevole economista, intervenendo su un importante quotidiano nazionale, lo ha addirittura indicato come uno degli elementi di possibile verifica della volontà riformatrice del Governo. Sono partito da questo punto perché voglio preliminarmente fare un'osservazione. Stiamo discutendo di un atto molto importante, non solo perché si fissano i saldi di finanza pubblica a cui poi la manovra di bilancio dovrà attenersi, perché questo DPEF traccia il programma della legislatura: è la prima volta che capita. Noi, la maggioranza (e sottolineo con qualche enfasi questa mia prima riflessione,

Nel programma della coalizione con cui ci siamo presentati agli elettori abbiamo posto la politica economica come elemento centrale della nostra proposta al Paese. anche attraverso questo Documento di programmazione, il programma politico diventa contenuto dell'azione di Governo. Quindi stiamo discutendo di un atto importante, non secondario, significativo

vogliamo che sia chiara la nostra analisi della situazione italiana. Mi diffonderò un po' su questo aspetto:

In una situazione in cui la difficoltà di crescita e l'insufficiente dinamismo economico costituiscono uno dei problemi dell'area dell'euro, e dell'Europa in generale, siamo cresciuti meno della metà di quanto è cresciuta l'Europa e l'area dell'euro.

in cui sono evidenti segni di dinamismo anche nell'economia italiana: lo hanno rilevato l'ISTAT e tutti gli istituti, anche di analisi congiunturale, auditi dalle Commissioni bilancio della Camera e del Senato nei lavori di preparazione del Documento di programmazione economico‑finanziaria. Nonostante questo dinamismo dell'economia italiana, la questione rimane aperta, perché permane il divario - che ho ricordato in precedenza - con gli altri Paesi. La Commissione europea prevede che nel 2006 il prodotto interno lordo italiano crescerà dell'1,3 per cento, un po' meno di quello che - ne parleremo il nostro Documento di programmazione, e che il prodotto interno lordo medio dell'area dell'euro crescerà del 2,1 per cento: dunque, quasi un punto in più. Nonostante un certo miglioramento della situazione, continuiamo a registrare questa differenza che rappresenta uno dei nostri più gravi problemi.

come diretta conseguenza dell'insufficiente capacità di crescita della produttività del nostro sistema economico. Il secondo problema dell'Italia è quello della crisi della finanza pubblica. Il Governo ha varato, all'indomani del suo insediamento, un'operazione verità; non ha rilasciato interviste al telegiornale della sera, come è accaduto nel 2001, ma ha insediato una Commissione per fare una vera e propria *due diligence* dei nostri conti. Secondo i risultati del lavoro della cosiddetta commissione Faini, l'aggiornamento del tendenziale di finanza pubblica comporta una stima al rialzo del rapporto tra *deficit* e prodotto interno lordo,

Il Documento sostiene anche che bisogna calcolare mezzo punto in più, derivato dai rischi della difficile attuazione dell'ultima manovra, sia sul piano della sua efficacia - ci ricorda la relazione - sia sul piano della sua capacità di realizzazione.

bilancio, di assumersi la responsabilità dell'attuazione di provvedimenti anche non condivisi della precedente manovra di bilancio. Di fronte a questi dati, l'opposizione in genere ha reagito non è molto, che in fondo si tratta soltanto dello zero e qualcosa, che il riferimento al 1992 come anno al quale assimilare la situazione dei conti pubblici del nostro Paese di quest'anno è un allarme ingiustificato.

Essi sanno bene che il problema principale a cui noi dobbiamo fare riferimento non è tanto l'indebitamento, cioè il rapporto tra il *deficit* e il prodotto interno lordo,

Negli ultimi tre anni il debito pubblico è di nuovo aumentato dopo una fase di progressiva, sia pure lenta, ma costante diminuzione.

crescita, risanamento, equità. Ciò vuol dire, cari colleghi, che nell'impostazione del Documento di programmazione economico-finanziaria del Governo e della sua maggioranza non esiste una politica dei due tempi. È necessario tornare a unire le azioni sul versante delle politiche di sviluppo alle azioni sul versante del risanamento dei conti, oltre che a quelle sul versante dell'equilibrio sociale. Questi tre temi sono tra loro strettamente collegati. Sono obiettivi legati tra di loro perché la crescita è indispensabile per produrre ricchezza e, se non si crea ricchezza e non si risanano i conti, non ci sono risorse da redistribuire. Il risanamento è necessario per consentire alla pubblica amministrazione di attuare politiche di sviluppo e di rafforzare le politiche di tutela dei ceti più deboli. L'equità è necessaria per realizzare l'equilibrio sociale e costruire un ambiente sociale favorevole allo sviluppo.

che abbiamo in mente è una strategia che leghi insieme obiettivi diversi e contribuisca a rendere possibile la costruzione di politiche di sviluppo compatibili con una società più equilibrata e più giusta. Entrambi questi obiettivi sono presenti nel DNA della nostra coalizione e delle strategie della nostra maggioranza. Attraverso quali strumenti il Documento di programmazione economico-finanziaria punta a realizzare una politica di crescita, di risanamento e di equità? Naturalmente, per l'approfondimento dei singoli punti rinvio alla relazione scritta, perché non potrei adesso

Per quel che riguarda le politiche di sviluppo, sottolineo il fatto che questo Documento di programmazione economico-finanziaria dopo molti anni imposta una strategia di politica economica basata sull'offerta, cioè sulla crescita della capacità competitiva del nostro sistema produttivo. La politica industriale era al centro del nostro programma di Governo; ora la politica industriale è al centro del Documento di programmazione. Riqualificazione del sistema produttivo, dimensione delle imprese, specializzazione settoriale, innovazione e ricerca, internazionalizzazione, riferimento alla Strategia di Lisbona come quadro generale per queste azioni: sono i contenuti di una moderna politica industriale che individuiamo come necessaria per rafforzare la capacità competitiva e di innovazione, la capacità da parte del nostro sistema produttivo

ed urgente: la riduzione del cuneo fiscale. Una riduzione che avvenga attraverso criteri selettivi, legati alla riqualificazione del mercato del lavoro, quindi privilegiando le imprese che puntano a creare occupazione di qualità,

Uno strumento che ha certamente il significato congiunturale di affrontare, prendendo il toro per le corna, il problema del costo del lavoro, ma che assolve al compito di preparare le strategie strutturali che ho già evidenziato.

nella giornata di ieri. C'è una strategia di apertura dei mercati, un elenco delle aree e dei settori in cui occorre intervenire e c'è la consapevolezza che riforme che non costano, capaci di rendere la società italiana più dinamica, più moderna e competitiva, in cui le risorse e le energie, soprattutto dei giovani, si possano sviluppare meglio, sono un potente strumento di crescita economica e di competitività.

è quella di riportare l'avanzo primario a livelli elevati. L'obiettivo è il 4,9 per cento nel 2011, riguardo, che esisteva un impegno informale assunto dall'Italia in sede europea, che era quello di mantenere in modo significativamente elevato l'avanzo primario per riconfermare la volontà e la capacità di una progressiva riduzione del debito pubblico.

e di aumentare l'efficienza. All'interno di tali settori esiste un grave problema di efficienza. Contemporaneamente, vi è un problema di contributo che questi settori devono dare alla riduzione della spesa.

ma sui saldi e sulla cooperazione nella definizione e nel raggiungimento degli obiettivi tra il Governo centrale e il sistema delle autonomie locali, un segno di riforma.

il Mezzogiorno continua ad essere quello che era nel nostro programma: una grande risorsa per il Paese che ha bisogno di investimenti, di crescita, di diventare il punto di riferimento della capacità dell'Italia di proiettarsi sui grandi scenari mondiali che, attraverso il Mediterraneo, ricollocano l'organizzazione geopolitica del mondo in termini diversi rispetto a quelli che siamo abituati a conoscere. Concludo con tre rapidissime

È un DPEF moderno: liberalizzazioni, concorrenza, società nuova, società aperta sono strumenti di crescita e di sviluppo. È un Documento che vede nella partecipazione uno dei punti fondamentali. Non a caso è scritto la definizione precisa degli strumenti da raggiungere la individueremo nella legge finanziaria perché le politiche specifiche devono essere il frutto della concertazione; una concertazione

ma a nostro parere non ha potuto illustrare i contenuti, visti i silenzi che fanno seguito a quei titoli nel contenuto del

Credo invece di dover condividere l'opinione espressa nelle audizioni, anche da parte del Governatore della Banca d'Italia: è utile il DPEF perché dà un quadro di coerenza per la politica economica. Giustamente il collega Morgando ha sottolineato che, come è avvenuto all'inizio della passata legislatura, della legislatura dà un quadro che va al di là dell'obbligo di legge triennale e riguarda il quinquennio dell'intera legislatura. Ciò detto, però, mi sembra di dover sottolineare subito, come ha accennato questa mattina in audizione il vice ministro Visco, che normalmente questi Documenti, almeno per l'80 cento, si assomigliano, da un passaggio all'altro delle maggioranze di Governo, perché in gran parte sono fatti dagli uffici interni, dagli uffici studi.

Non è un documento sulla politica economica; per di più, un documento da centro studi carente dal punto di vista dell'analisi economica, per alcuni aspetti che sottolineerò, totalmente carente in termini di indicazioni di politica economica, di strategia. vero infatti che a settembre discuteremo il disegno di legge finanziaria, che incarnerà quella strategia, ma è altrettanto vero che è opportuno che nel mese di luglio si definisca il quadro strategico della politica economica. Ebbene, al di là dei titoli che il collega Morgando ha passato in rassegna, il Documento eccelle per un gravissimo silenzio che, a detta dei tecnici che hanno probabilmente stilato il Documento, potrei definire esogeno: un silenzio totale che riguarda l'andamento dell'economia mondiale ed europea, che rappresenta il quadro di riferimento dal quale dipendono i tre quarti di qualunque risultato economico del nostro Paese. Nel Documento si evidenziano anche due silenzi endogeni, riferiti al rapporto tra Italia ed Europa e a quello tra Italia e Italia.

Qual è il ruolo dell'Italia e dell'Europa nel governo mondiale dell'economia? Ci rendiamo conto che l'economia mondiale è dominata, sul piano della crescita reale, da quello che qualcuno chiama l'asse del Pacifico, che lega Stati Uniti e Cina, e dalla scomparsa dell'asse Atlantico e, ancor peggio, dell'asse del Mediterraneo? Ci rendiamo conto che da sette-otto anni è cambiata l'era del mondo? Ci rendiamo conto che questo andamento dell'economia reale è totalmente insostenibile? Certo, si è invertito l'andamento delle ragioni di scambio che per quarant'anni ha consentito al ricco Nord del mondo

europeo e italiano negli ultimi quarant'anni, pagato in larga parte dalle risorse del Sud del mondo. Se consideriamo la media dei tassi di crescita del Nord America, dell'Europa e dell'Asia degli ultimi sette anni e la proiettiamo nel prossimo futuro, l'attuale G8, tenutosi pochi giorni fa con la presidenza russa a San Pietroburgo,

ma il silenzio del DPEF è sul nodo della crescita dell'Europa continentale, con in testa Germania, Francia e Italia, e non è questione da poco. Su tale sfondo di squilibrio dell'economia reale, è un continente perduto, l'Atlantide del Terzo millennio. Si tratta dell'Africa, che, in tale quadro, nel giro di cinque o dieci anni, porterà a bussare alle nostre porte 50 o 60 milioni di esseri umani: ci saranno, forse, né leggi, né mitra per impedire tale afflusso incontrollato e incontrollabile. L'Italia, che è al centro del Mediterraneo,

dal punto di vista geopolitico, possiamo parlare di una *governance* internazionale con una potenza economica e politica come la Cina, che tiene con il cappio al collo l'altra grande potenza del mondo, gli Stati Uniti, possedendo il 50 per cento del suo debito estero.

Ma, cari colleghi, sapete qual è la conseguenza di quella riga? Stiamo predeterminando *ex ante* un totale silenzio italiano in ambito europeo, un totale silenzio europeo in ambito della *governance* mondiale, che portano via due punti di crescita l'anno di PIL per tutta l'Europa continentale. Poi discutiamo delle politiche dell'offerta, sacrosante, delle politiche industriali, sacrosante, ma quel mezzo punto di differenza tra la media della crescita italiana e la media della crescita europea è ben poca cosa se non visto e inquadrato nei due punti che rinunciamo *ex ante* ad avere perché non svolgiamo un ruolo politico in Europa e non svolgiamo un ruolo politico, con l'Europa, nel resto del mondo. Quindi, politica monetaria assegnata alla Banca centrale europea; politica di bilancio assegnata al Patto di stabilità e crescita, nel quale la parola «crescita» è stata cancellata:

Dopo di che, come abbiamo fatto nei giorni scorsi, litighiamo tra maggioranza e opposizione se c'è da mettere l'etichetta del pane fresco o del pane conservato nella nostra distribuzione commerciale; cosa importante, ma francamente ritengo che una riflessione su questi temi debba trovare luogo e momento seri per essere fatta. Questo è il silenzio esogeno

c'è un altro silenzio endogeno. Il collega Morgando e il presidente Morando in Commissione hanno detto che il DPEF indica con chiarezza le linee di intervento. anche ricordato che i capitoli più imponenti della spesa pubblica sono pensioni, sanità, pubblico impiego ed enti locali.

perché all'interno di ciascuno di questi settori ci sono gli stipendi, gli acquisti, le consulenze, tutte le voci economiche di classificazione della spesa.

cosa dire della spesa per acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione? Cosa dire dello strumento CONSIP

ha ragione l'attuale maggioranza: è vero, nella passata legislatura la spesa corrente è cresciuta. Ma debbo ricordare che in queste Aule parlamentari una strana alleanza trasversale si è opposta all'opera di contenimento di quella spesa. Nulla a che vedere con la salute, salute, nulla a che vedere con gli stipendi, bensì mille rivoli di rendite di posizione che, all'interno di quella spesa, determinano, non sani profitti di impresa, ma rendite dovute ad incrostazioni forse ultradecennali. Cosa dire dei 13 miliardi di euro che ogni anno il Parlamento assegna in conto capitale ai fondi perduti? Quale efficacia ed efficienza di queste tasse dei contribuenti spostate nelle tasche di alcune iniziative, che forse dopo qualche anno, di perduto hanno proprio le iniziative, oltre che i fondi? Cosa dire dei 16 miliardi di contributi in conto corrente a tutte le imprese? 29 miliardi all'anno di tasse dei contribuenti spostati in queste due voci di spesa, sulle cui capacità

dei dati contenuti nello stesso DPEF. A fronte di questa indicazione di politica economica, tra gli obiettivi posti dal Governo per Governo per l'anno prossimo c'è un freno alla crescita economica, ovviamente come contropartita del contenimento del *deficit* pubblico.

interno lordo in più dopo cinque anni, alla fine di una legislatura, e comunque sempre lontano da quanto accade nel resto d'Europa e del mondo. Allora, la sintesi politica è che c'è una scelta politica chiara. di un problema di prudenza, ma di supina acquiescenza agli interessi finanziari dell'Europa e dell'Italia. Certamente il risanamento finanziario è cosa buona e giusta, ma non può esaurire

che addirittura, all'interno di una maggioranza che, ripeto, si definisce di centro-sinistra con questi obiettivi, vi sia una sinistra chiamata radicale, più spinta (almeno a parole) sul sociale,

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghe senatrici e colleghi senatori, il senatore Morgando ha illustrato in modo molto puntuale e preciso i contenuti del Documento esame e ha abbozzato anche i lineamenti della risoluzione conclusiva che la maggioranza proporrà. Ho ascoltato con molta attenzione anche l'intervento del relatore di minoranza, senatore Baldassarri, il quale mi pare abbia sostenuto che con questo la maggioranza ed il Governo rinunciano all'obiettivo della crescita per il prossimo quinquennio e sarebbero - utilizzo le parole del senatore Baldassarri - prigionieri dei grandi poteri finanziari. Ora, francamente non capisco questa critica che viene dal rappresentante di una parte politica che ha avuto nella scorsa legislatura delle precise responsabilità di Governo (il senatore Baldassarri era vice ministro all'economia) e che ha prodotto attraverso una politica economica e finanziaria fallimentare - questo non è un giudizio di valore, ma un giudizio tecnico sulla base dei dati a disposizione - una diminuzione del tasso di crescita del nostro Paese.

di questo genere; mi sto riferendo al suo intervento in cui lei ha detto che il DPEF non considera abbastanza l'obiettivo della crescita e al fatto che negli ultimi cinque anni la crescita, nonostante fosse costantemente sovradimensionata nelle vostre finanziarie, anche per sovradimensionare le entrate,

di crescita economica strettamente correlati agli altri obiettivi del risanamento e dell'equità, lo considero assolutamente giusto e indispensabile per rimettere ordine innanzi tutto

obiettivi di crescita realistici ma costanti, mettendo contemporaneamente mano a quel risanamento delle finanze pubbliche che è assolutamente indispensabile. Anche qui, senza alcuna polemica, basta citare alcuni dati:

di potere finanziario o economico, semplicemente c'è la volontà di ricollocare l'Italia, la sua economia e la sua finanza pubblica nell'unico contesto in cui può crescere e svilupparsi, quello europeo. Anche qui c'è una visibile correzione rispetto all'antieuropeismo al quale era improntata la vostra politica economica e di Governo. Vengo adesso a un piccolo giallo che è esploso, se non sbaglio, negli interventi preliminari a questa discussione, a proposito del parere della la Commissione affari costituzionali.

della spesa pubblica italiana passa attraverso le Regioni e le autonomie locali e il 64 per cento - sono dati recenti - degli investimenti dell'intero sistema delle pubbliche amministrazioni è effettuato dal sistema delle Regioni e delle autonomie locali. Occorre quindi invertire la tendenza che negli ultimi cinque anni è nettamente prevalsa a decidere misure di contenimento, di tetti, di costrizioni, che alla fine hanno prodotto due risultati inequivocabili: da un lato, la spesa anziché diminuire è complessivamente aumentata - questo ci dicono gli indicatori - e dall'altro, si sono compresse le potenzialità di contributo del sistema delle Regioni e delle autonomie locali alla crescita del Paese. Come vede, senatore Baldassarri, anche a me interessa molto il tema della crescita, tant'é che sottolineo un punto importante contenuto nel DPEF: si vuole ridare senso al Patto di stabilità interno trasformandolo, come in Europa, in un Patto di stabilità e crescita. Secondo me questo è essenziale perché occorre corresponsabilizzare il sistema delle Regioni e delle autonomie locali sui grandi obiettivi di finanza pubblica, non solo non solo sul versante del contenimento che in alcuni casi è necessario, ma anche come fattori fondamentali di sviluppo del Paese. In questo contesto si può utilizzare una grandissima risorsa per il risanamento delle casse pubbliche, ma anche per la crescita del Paese, che si chiama autonomia,

ancora in gran parte centralizzato. Occorre dare equilibrio a questi due fattori in modo tale che sia possibile, anche in questo caso, cogliere il grande fattore positivo di un sistema finalmente di accordi, di patti, di concertazioni tra Regioni, enti locali e Stato che sostituisca quella guerra permanente, quel conflitto istituzionale permanente, che in questi cinque anni ha prodotto gravi danni sia per la crescita del Paese che per i parametri fondamentali di finanza pubblica. È assolutamente discutibile il fatto che la stessa fosse in distribuzione perché chi l'ha letta, chi l'ha presa, poteva anche pensare che fosse stata approvata e non fosse solo, appunto, una bozza. È iscritto a parlare il senatore Cutrufo. Ne ha facoltà. Signor Presidente, il ministro Padoa-Schioppa ha affermato che sono necessarie robuste correzioni dei conti nei prossimi due-tre anni, tali da ricostituire un *surplus* primario sufficiente a garantire la sostenibilità del bilancio pubblico e la riduzione del debito. Sarebbero necessarie, quindi, delle misure correttive strutturali che consentano di abbandonare quelle che lo stesso ha definito «politiche di interventi *una* *tantum,* che hanno finora portato benefici temporanei». ci lascia, tuttavia, alquanto perplessi, almeno dopo aver preso atto del testo del DPEF proposto. Infatti, ad un attento osservatore non può in alcun modo sfuggire l'evidenza, e cioè che l'intero Documento non contiene scelte di natura realmente strategica, sotto molti profili, invece, necessarie per il nostro Paese. Molte parti del Documento, soprattutto in settori chiave della nostra economia, risultano lacunose, eccessivamente generiche e prive di sostanziale fondamento. Ancora una volta, il Governo si è mostrato difficile ad operare un reale confronto con le categorie interessate. Viva la concertazione, si potrebbe dire, ma essa non è stata la nostra bandiera - ancorché sia tra le nostre convinzioni - in campagna elettorale. La quasi totale assenza di misure concrete volte al risanamento della finanza pubblica, così compromessa per affermazione del solo Governo, è indice chiaro di una tendenza perversa verso la quale la sinistra si è avviata. Numerose sono le critiche emerse durante l'esame del Documento da parte dei componenti le Commissioni preposte all'esame. Sicuramente la nota più preoccupante è la prospettiva di tagli alle spese sociali: pensioni, sanità, enti locali; sono le maggiori sigle sindacali a lanciare un grido di allarme poiché, inevitabilmente, la compressione della spesa sociale inciderà negativamente sui servizi resi ai cittadini. Contestualmente, sono del tutto assenti indicazioni circa la linea che la maggioranza intende perseguire in tali settori. Si cerca così di perseguire l'ambizioso obiettivo, più volte millantato, del risanamento dei conti pubblici, ma si prescinde totalmente dal prevedere un corretto sostegno allo sviluppo economico, incentivi agli investimenti e riduzioni delle spese di parte corrente. Vengono inoltre indicati tempi irrealisticamente brevi, soprattutto se non accompagnati dalla previsione di nuove entrate fiscali, se non quelle determinate dalla lotta all'evasione, che restano ancora virtuali, finché non realizzate, il che ci porta a temere un preoccupante scenario in cui potranno essere colpite le pensioni, la sanità, gli enti locali, il pubblico impiego. Sarebbe invece stato necessario prevedere almeno un anno in più nella manovra di rientro, permettendo così un approccio più morbido e diluito, il quale non comprometterebbe la prospettiva di rientro nei parametri e non finirebbe con il pregiudicare la ripresa economica del Paese, che potrebbe essere invece negativamente condizionata da una manovra così pesante e così congegnata. Infatti, invece di puntare ad una concreta forma di stabilizzazione del rapporto tra debito e PIL e di concedere almeno un anno in più di tempo per programmare il rientro nei parametri previsti dai Trattati europei, la prevista manovra di rientro del *deficit* costringerà il Governo ad una finanziaria di 35 miliardi di euro che porterà inevitabilmente con sé tagli alla spesa sociale e una ferrea stretta sugli enti locali. Al tanto decantato lavoro di tipo analitico riguardo la situazione corrente del Paese non è seguita un'altrettanto concreta definizione delle misure da adottare per il raggiungimento degli obiettivi, che troppo spesso rimangono solo degli enunciati di principio. Manca qualsiasi scommessa su forme di politica economica e finanziaria nuove. La ricetta sulla politica delle entrate è quella più tradizionale: tagliare la spesa pubblica e in modo specifico, appunto, pensioni, sanità ed autonomie locali. Sicuramente potrebbe essere degno di nota l'impegno nella lotta all'evasione fiscale,

il merito dei quali, naturalmente, deve essere riconosciuto al precedente Governo. Ma tali risultati positivi sono stati il frutto di una strategia complessiva messa in atto da una maggioranza coesa e compatta, qualità che non può di certo rinvenirsi oggi nell'attuale maggioranza. Un Documento così congegnato sembra, a noi del Gruppo Democrazia Cristiana-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia, totalmente incapace di favorire qualsiasi forma di rilancio economico del nostro Paese, analogamente a quanto è accaduto con il decreto-legge Le logiche proposte sono spesso superate ed irrealistiche, prive di concrete indicazioni sull'utilizzo delle risorse finanziarie necessarie al risanamento dei conti pubblici. Così, critiche sono le previsioni in tema di infrastrutture, ove vi è anche una evidente elusione della legge obiettivo, che impone al Governo di presentare l'allegato infrastrutture, il quale deve dare precisa indicazione sulle priorità in concomitanza con la presentazione del DPEF. Tale allegato invece risulta alquanto generico e non contiene alcuna previsione di natura programmatica. Poco condivisibile è anche la logica con la quale è stata fissata la nuova gerarchia delle priorità, la quale viene fatta dipendere da un mero stato di avanzamento che esclude qualsiasi pianificazione o confronto con le realtà locali coinvolte e soprattutto non tiene conto delle specifiche necessità del Mezzogiorno. Sentendo il relatore, peraltro, questa speranza l'abbiamo; staremo a valutare i fatti, e da ciò che abbiamo visto in questi sessanta giorni tanta speranza in verità non l'abbiamo. Tutto ciò, poi, a dimostrazione di un sottinteso avallo della politica in materia posta in essere dal Governo di centro-destra e tanto criticata in sede elettorale, anche attraverso la riconferma delle risorse già stanziate nella precedente legislatura, paradossalmente invece criticate negli anni passati, specialmente durante la campagna elettorale. Lo stato dei fatti avalla la nostra opinione che l'attuale Governo manchi di proprie linee programmatiche anche nel settore delle infrastrutture, soprattutto in comparti attualmente nevralgici i quali chiedono un incisivo intervento, come quello dell'Alta velocità, soprattutto nel Meridione, e nel settore portuale, per non parlare poi dell'araba fenice, che per noi era concretezza, del ponte sullo Stretto di Messina. Ed ancora. Si fa positivamente riferimento all'applicazione del Trattato di Kyoto, ma non sono evidenziati o predisposti gli strumenti per rendere concretamente operativo questo orientamento. O nel settore della difesa, ove il Documento continua a rimanere pieno di indicazioni generiche, come il richiamo ad uno «snellimento dell'amministrazione». O in tema di politiche fiscali, ove mancano i riferimenti alle spese di investimento o la valutazione degli effetti di un'ampia riduzione del prelievo fiscale. Vi è anche da sottolineare la riduzione delle risorse disponibili per la politica estera, senza tuttavia prevedere alcuna forma o volontà di procedere ad una concreta razionalizzazione delle strutture del Ministero degli affari esteri o ad un adeguamento delle strutture diplomatiche e consolari agli attuali impegni internazionali. Positivo potrebbe invece essere il riferimento alla necessità di puntare alle fonti rinnovabili di energia, ma bisognerà capire come tradurre tutto ciò in impegni realmente concreti nella prossima finanziaria. Critico è l'intervento riservato al terzo settore, che anziché essere considerato nella sua insita capacità di apportare una crescita nelle relazioni di solidarietà del Paese è divenuto un mero strumento di supporto per coprire tutte quelle necessità cui, a causa dei tagli, lo Stato non sarà in grado di provvedere. Nel Documento si fa una sorta di presa d'atto della situazione drammatica in cui versano la ricerca e l'innovazione in Italia ma, come al solito, in concreto mancano chiare ed incisive strategie di rilancio dell'intero sistema formativo ed universitario oltre che di quello, fondamentale, di incentivi alla ricerca. Paradossale poi è il fatto che si ritiene possibile effettuare interventi a costo zero ed un impegno finanziario è ritenuto solo "auspicabile", non necessario. non necessario. Non vi sono linee di indirizzo o impegni precisi in tema di politiche pubbliche in materia di lotta alla povertà e di aiuto pubblico allo sviluppo. Non vi è nemmeno alcun cenno alla posizione e al peso del nostro Paese di fronte agli obiettivi assunti in sede internazionale nell'ambito delle Nazioni Unite. Anzi, sono stati ridotti i contributi versati dall'Italia alle agenzie delle Nazioni Unite come l'UNICEF. Molti altri sarebbero i rilievi critici da muovere a questo primo Documento di programmazione economica dell'attuale maggioranza, specialmente alla luce della feroce campagna elettorale effettuata, che ha portato ad una demonizzazione dell'operato del Governo di centro-destra soprattutto in tema di conti pubblici. Ai buoni intenti dichiarati, in ambito di strategia economica, da questo Governo, sono solo seguiti interventi poco concreti, di scarsa qualità e poco coerenti con il preannunciato programma di Governo. Con rammarico per il nostro Paese, noi del Gruppo Democrazia Cristiana-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia non possiamo in alcun modo condividere l'operato messo in campo con questo DPEF dall'attuale maggioranza ed auspichiamo una maggiore incisività e concretezza nelle successive fasi della manovra.

finora sentito (basta leggere i giornali di oggi) vi è una valutazione da parte di economisti, i più disparati, non di una opacità o di un riduzionismo di questo Documento sul quale stiamo conducendo una pacata discussione, ma al limite, paradossalmente, di un eccesso di ambizione strategica che pure si dilata in un quinquennio, quindi su un periodo vasto, ma di cui, come dire, si coglie, si apprezza, lo sforzo, lo spirito, la latitudine strategica. Diversamente da quanto affermato dal senatore Baldassarri, non è affatto vero - almeno questa è la mia sensazione - che il DPEF taccia sugli scenari internazionali. Anzi, ad essi è dedicata tutta la prima parte. Forse, la conseguenza e la sintesi politica che se ne trae (certo non in

dei rischi, per ciò che riguarda la ricaduta sulla situazione italiana, riferiti agli squilibri finanziari globali, al rischio di un forte e disordinato indebolimento del dollaro, al rialzo del prezzo del petrolio, alla possibilità di una caduta degli elevatissimi

e monetaria europea o che - come sembrava aver dedotto indirettamente il senatore Baldassarri - l'area europea non debba proporsi come grande soggetto finanziario ed economico integrato con una sfida globale.

relativa libertà intellettuale che ci è dovuta e che si può esercitare quando si parla dell'interesse nazionale e dell'emergenza nazionale.

il senso di questo DPEF: è un documento a cui sarà ancorata non un'inutile esercitazione letteraria o politologica, ma che impegnerà il Governo e la volontà parlamentare per una previsione e una prescrizione di saldi. Quindi un documento sul quale il Parlamento, finalmente fuori dalle strettoie dei voti di fiducia, può esercitare la sua analisi, il suo confronto, la sua sfida

misurarsi non sull'angusto e stretto lasso di una legislatura, ma sugli ultimi dodici anni. Non importa, pertanto, quali legislature si siano succedute, quali fasi politiche e quali congiunture mondiali.

al peso dell'economia della conoscenza e dell'investimento nella ricerca e nella scuola, così efficacemente sottolineato nel DPEF, e alla prospettazione di nuovi assetti tra economia, università territorio, che possono far sperare che, anche attraverso l'investimento nella ricerca e nella scuola, si sviluppi e tragga forza un fattore nuovo di competitività locale e nazionale

Nel 2001 le parole d'ordine che sostanziavano quel documento erano "meno tasse" e "meno spesa corrente". Nel 2006 la scommessa è di realizzare più crescita, più risanamento, più equità. Devo dire subito che, secondo me (poi sono i numeri a dimostrarlo),

sul sistema pensionistico, sul pubblico impiego, sul servizio sanitario, sulla finanza degli enti decentrati.

essenziali garantiti dall'intervento pubblico. Avremo la possibilità, nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, di sviluppare il confronto, anche attraverso una politica di concertazione, su

di scegliere quando andare in pensione. Sarà una questione sulla quale il confronto dovrà svilupparsi in modo molto rigoroso. Ritengo sia corretto intervenire sul sistema della pubblica amministrazione con obiettivi di stabilizzazione del precariato e, soprattutto, di sostituzione del *turn over*, ringiovanendo così la forza lavoro all'interno della

che definisco "autocentrato". Il Protocollo di Kyoto è visto come una grande opportunità per rinnovare il nostro sistema, per renderlo più efficiente, per impostare politiche di risparmio energetico, per ridurre gli sprechi

La manovra ovviamente è complicata e molto rilevante dal punto di vista dell'ammontare.

rispetto a quanto previsto per il 2007; però se già nel 2007 impostiamo le misure probabilmente sul piano strutturale avremo effetti anche negli anni successivi. Da questo punto di vista, potrebbe trattarsi di una manovra più sostenibile.

della sua stabilizzazione. In questo modo ci potrebbero essere più risorse da destinare allo sviluppo, ai settori sociali e e ad obiettivi di contenimento e di sostenibilità per la società nel suo complesso. Se l'obiettivo è quello di tenere insieme crescita, risanamento e sviluppo,

Signor Presidente, colleghi senatori, oggi ho sentito sia il relatore sia i colleghi di maggioranza citare

possibile disponibilità già dalla prossima legge finanziaria. La legge finanziaria per il 2007 - dice il Documento - disporrà interventi, il cui importo complessivo viene quantificato in circa 20 miliardi di euro al netto di nuove spese, volti

il Documento di programmazione economico-finanziaria non individua soluzioni concrete per raggiungere gli obiettivi che si prefigge: parla di crescita, risanamento ed equità, come abbiamo sentito più volte e come è esplicitamente indicato.

Il risanamento è altrettanto importante, perché fa leva, naturalmente, sulla necessità di controllare la spesa corrente, che crea le difficoltà di finanza.

indicato sotto il profilo fiscale nel decreto Bersani, procedendo in quella direzione. Se infatti equità vuol dire continuare ad irrigidire il controllo e il prelievo nelle aree che già

Tra parentesi, nel DPEF - a proposito di crescita, sviluppo ed equità - viene precisato che, come ho ricordato poc'anzi, uno dei problemi fondamentali è proprio il controllo della spesa pubblica corrente. Se la politica delle entrate

non capiamo perché l'Esecutivo non abbia anticipato provvedimenti puntuali e dettagliati, rinviando, invece, il momento decisionale il più a lungo possibile nell'ambito della manovra di bilancio.

Basti pensare ad una delle misure più rilevanti annunciate dal Governo in materia di taglio del cuneo fiscale, a beneficio sia delle imprese, sia dei lavoratori, in modo da stimolare contemporaneamente investimenti e consumi. Non è del tutto scontato che tale misura porti i risultati previsti dal presidente Prodi, sia perché gli effetti degli sgravi rischiano di andare a beneficio delle produzioni a più alta intensità di lavoro (piuttosto che a quelle a più alto contenuto tecnologico), sia perché non è sicuro che lo sgravio venga utilizzato dalle imprese per ridurre i prezzi dei prodotti (piuttosto che per aumentare i margini di profitto). Non si stabilisce, inoltre, se esso sarà a carattere selettivo o generale, con l'ulteriore rischio di una polverizzazione dei benefici. In tali condizioni, non si comprende come tale misura possa avere effetti concreti in termini di aumento della produttività e della competitività del sistema, senza risolversi, piuttosto, in un intervento simbolico molto costoso ma sostanzialmente inutile.

vi sarà una maggioranza compatta a sostenere quest'ultima, o vi saranno le resistenze di Rifondazione Comunista, che ha già manifestato, nelle Commissioni, posizioni di dissenso sia sul testo del Documento in esame, sia sul tempi del piano di rientro del disavanzo concordati in sede di Unione Europea, considerati troppo ristretti?

Le misure dovrebbero essere dirette a contenere la spesa previdenziale (con l'innalzamento dell'età pensionabile), a prevedere nell'ambito della pubblica amministrazione determinati meccanismi e a tagliare gli sprechi nel settore della spesa pubblica, in particolare quello sanitario. Sappiamo bene che i settori in cui si verifica maggiormente lo scostamento rispetto alle previsioni di spesa sono proprio la sanità e gli enti locali, che non sono sotto il diretto controllo dello Stato, ma che gravano pesantemente sul bilancio pubblico. Per cui è condivisibile l'introduzione della politica dei saldi piuttosto che di quella del tetto massimo, ma sarebbe necessario introdurre, nell'ambito della finanza decentrata, il principio di responsabilità della spesa, interrompendo il flusso continuo e incontrollabile di trasferimenti. Tutti, a livello sia decentrato sia di amministrazione centrale, devono essere chiamati a comportamenti responsabili, premiando quelli virtuosi e penalizzando gli sprechi, con l'introduzione di un efficace controllo di gestione. A proposito dell'equità fiscale del sistema, di cui pure si parla diffusamente nel Documento di programmazione economico-finanziaria, è necessario rispettare il principio di progressività così come stabilito in Costituzione. In tema di lotta all'evasione sarebbe poi opportuno prevedere meccanismi basati sul contrasto di interessi. Questi sono solo alcuni dei temi che andrebbero affrontati, ma prima ancora andrebbe posto un interrogativo di fondo: di cosa ha bisogno il Paese? La prima risposta è sicuramente di liberalizzazioni, che però non tocchino solo aspetti marginali, come nel caso del provvedimento approvato ieri, ma che coinvolgano settori essenziali per l'intero sistema produttivo, primo fra tutti quello dell'energia, in cui sono necessari investimenti per costruire nuovi impianti al fine di diversificare fonti e fornitori e calmierare il costo energetico. Sarebbe poi necessario incrementare e innovare la rete infrastrutturale, logistica e dei trasporti, che costituisce il ganglio vitale per rilanciare lo sviluppo e la crescita del sistema produttivo e, soprattutto, la sua capacità di competere. Su questi temi non esiste, a nostro parere, una questione settentrionale o meridionale, poiché è l'intero sistema Paese che deve affrontare nuove sfide generate dalla globalizzazione e dalle profonde trasformazioni sociali ed economiche a livello internazionale. Sullo scenario mondiale si sono affacciati prepotentemente nuovi soggetti "affamati", che sono diventati dei *competitor* temibili che utilizzano il *dumping* sociale e ambientale per conquistare fette sempre più ampie di mercato. Di fronte ad essi l'Italia appare un Paese sazio, che ha bisogno di trovare la strada di una crescita che non derivi da fattori contingenti ed esterni, ma che nasca da mutamenti strutturali dell'intero sistema. Non c'è possibilità di ripresa senza che vengano affrontati e risolti alcuni nodi fondamentali: in primo luogo, la tenuta dei conti pubblici, con l'attuazione di politiche di contenimento della spesa, soprattutto della pubblica amministrazione, il cui apparato dovrebbe essere snellito privilegiando la qualità e il risultato e non la quantità; in secondo luogo, la razionalizzazione del sistema delle entrate, che condurrebbe ad un miglioramento del rapporto *deficit*-PIL; infine, ma non meno importante, l'attuazione di politiche di sviluppo e di sostegno delle imprese con incentivi all'innovazione tecnologica, alla ricerca e alla crescita dimensionale del sistema industriale, al fine di perseguire l'obiettivo principale: il recupero di competitività. Per affrontare e risolvere i problemi e le sfide del futuro occorre però avere la consapevolezza che la lunga fase di crisi attraversata negli ultimi decenni ha radici profonde ed investe non solo l'aspetto sociale, economico e politico. Si tratta prima ancora di una crisi culturale, quindi più grave, il cui superamento deve ripartire proprio dalla cultura. Occorre riappropriarsi di valori troppo a lungo mortificati dalla cultura del '68, basata sul concetto di un falso egualitarismo, che ha poi condotto sul piano sociale ed economico ad una diffusa deresponsabilizzazione ed ha giustificato l'adozione di politiche di svalutazione, con conseguente crescita abnorme del debito pubblico. Occorre quindi un netto cambiamento di rotta che rivaluti il merito, il rischio, la competizione e che incida sulla mentalità e sui comportamenti di tutti i soggetti coinvolti, pubblici, privati, consumatori. Sappiamo bene che si tratta di innovazioni profonde e difficili che hanno effetto nel medio e lungo periodo travalicando i cicli elettorali, ma sono questi i cambiamenti di cui l'Italia ha bisogno per uscire dall'*impasse* della crisi. C'è solo da chiedersi se la classe dirigente, sia politica che economica, e la grande e media borghesia del Paese abbiano la capacità, il coraggio e gli strumenti per intraprendere questa strada e operare scelte difficili quanto necessarie o se non si preferisca continuare con interventi contingenti, di facciata, inadeguati e non duraturi, come nel caso del Documento di programmazione economico-finanziaria presentato dal Governo.

favorisce quelli che il sistema economico mette in fondo alle gerarchie sociali. Il Documento presentato si può leggere anche come una bandiera issata sulla testa della gente,

di internazionalizzazione delle imprese e dell'investimento nei settori strategici con caratteristiche di innovazione di processo e di prodotto.

condizione di lavoro. Siamo stati abituati a pensare che le forme di caporalato che abbiamo conosciuto nel Mezzogiorno in agricoltura fossero un portato del Medioevo,

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la finalità del Documento di programmazione economico-finanziaria è evidentemente quella di tracciare le linee guida del futuro sviluppo economico del Paese.

del libro delle buone intenzioni e della sagra dell'ovvietà che caratterizza questo scarno Documento di programmazione economico-finanziaria si debba forse fare qualcosa di più. attenersi al vero andando a ricercare le interpretazioni autentiche di coloro che sono istituzionalmente preposti a dar corpo, sostanza e materia a quelle linea guida. Tracciando rapidamente un quadro di quanto emerso fino ad oggi proprio in tema di interpretazione autentica, credo sia opportuno intanto rileggere ciò che il DPEF afferma in tema di politica dell'energia. al fine di garantire la sicurezza delle forniture, l'Italia, come altri Paesi europei, dovrà promuovere la diversificazione delle fonti primarie e la realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento di gas naturali, quali terminali di GNL, gasdotti, stoccaggi in sotterraneo e altro. come questa, che mi sembra essere di per sé più che una buona intenzione, possa conciliarsi con una posizione assolutamente antitetica

Sempre nell'ambito di quelle due audizioni - parlo quindi di interpreti autentici, cioè di autorevoli membri di questo Governo - in materia di cosiddette fonti rinnovabili, al di là del manifesto ideologico di tipo ambientalista che abbiamo sentito declamare dal ministro Pecoraro Scanio, abbiamo avuto dal ministro Bersani un'indicazione di segno completamente contrario, cioè l'assoluta consapevolezza che il problema energetico non si affronta e non si risolve in alcun modo cercando, soltanto surrettiziamente, di parlare di fonti alternative. Questa è una prima inconciliabile divergenza che di per se già determina una paralisi dell'attività governativa in uno dei settori chiave, che è quello dell'energia. Affrontiamone un altro, sempre in rapida sintesi, che è quello delle infrastrutture perché, sempre attraverso le interpretazioni autentiche, dal Ministro delle politiche del territorio (che è sempre il ministro Pecoraro Scanio) ci siamo sentiti declamare un'altra petizione di principio, una contrarietà assoluta al sistema della legge obiettivo. Ciò mi porta a domandarmi come sia conciliabile questa posizione con quella espressa, sempre nel corso di un'audizione in 13ª Commissione, dal Ministro delle infrastrutture il quale ha detto esattamente il contrario,

Il ministro Di Pietro ci ha quindi detto esattamente il contrario di quello che ci ha detto il ministro Pecoraro Scanio: il punto di partenza dell'attività del suo Dicastero sarà proprio quel piano delle infrastrutture che il Governo Berlusconi aveva varato tra il 2001 e il 2006. posizione totalmente e completamente inconciliabile con quella espressa da altro Ministro - il Ministro delle politiche ambientali e del territorio - che, tra l'altro, ha già detto con grande chiarezza che intende interferire in ognuna delle politiche legate al territorio. al territorio. In questo Documento di programmazione economico‑finanziaria si individua, tra l'altro, quale strumento di rilancio della competitività del Paese, la cosiddetta valutazione ambientale strategica che viene legata ad un piano delle grandi opere, il quale evidentemente non potrà mai decollare nella misura stessa in cui oggi non c'è e mai vi sarà, visto che due dei Ministri che dovrebbero concorrere a formarlo hanno al riguardo una visione totalmente e completamente inconciliabile. Mi pare quindi che, anche sul piano infrastrutturale, al di là della novella delle buone intenzioni, poco o nulla vi sia contenuto. Andiamo però oltre: l'ambiente viene individuato nel Documento di programmazione economico-finanziaria come una delle altre risorse e, sempre volendosi attenere alle interpretazioni autentiche di coloro che questa manovra dovranno poi in concreto sviluppare (cioè i titolari dei relativi Dicasteri), Dicasteri), ci sentiamo dire, sempre dal ministro Pecoraro Scanio, che la linea fondante della sua attività sarà l'abolizione della delega ambientale. dato che stiamo parlando di sviluppo del sistema Paese, sarà forse opportuno illustrare ai colleghi che non fanno parte della 13ª Commissione che cosa ci è stato detto da tutto il sistema imprenditoriale - non soltanto dalla dottoressa Marcegaglia per Confindustria, ma anche dai rappresentanti di Confartigianato, della CNA e di tutte le altre categorie proprio in relazione a quello che sarebbe l'effetto della soppressione della legge di delega ambientale: un vuoto legislativo preoccupante, ma, soprattutto, un danno incalcolabile per il sistema produttivo del Paese e l'incapacità di competere di competere in una dimensione di carattere globale della competizione economica con gli altri Paesi. Da questo punto di vista abbiamo un elemento che non è soltanto di contraddittorietà tra Dicasteri, ma è anche di totale inconciliabilità tra ciò che la parte produttiva del Paese segnala e le intenzioni manifestate come uno dei presupposti fondanti - forse anzi quello più fondante - la futura azione di governo da parte del titolare del relativo Dicastero. Non possiamo pertanto dire che l'ambiente in questo caso diventa una risorsa e che questo Documento, così come concepito, darà qualcosa in termini di sviluppo. Ma vi è di più, onorevoli colleghi: proprio lo stesso ministro Pecoraro Scanio ha dovuto ammettere che fra il 2001 e il 2006 vi è stato un incremento del 17 per cento annuo nella frequentazione dei parchi, individuati come risorsa del territorio. Il Ministro si è però forse dimenticato di dire che, in realtà, tra il 2001 e il 2006 è completamente cambiata in questo Paese la logica di fruizione del territorio anche nelle aree protette, che non è più stata vista come una campana di vetro da calare sul territorio sterilizzando tutto quello che c'è al suo interno, magari facendolo gestire occasionalmente da qualche cooperativa rosso-verde, eliminando tutto ciò che si trova all'interno, ma è stata vissuta in una chiave completamente diversa. Guarda caso, una delle altre linee guida fondanti è proprio quella di una restaurazione del passato - ovvero la logica delle campane di vetro

visioni strategiche totalmente inconciliabili fra di loro e tali, proprio per la loro inconciliabilità, da annullarsi a vicenda, determinando fatalmente la paralisi del sistema Paese. Una maggioranza senza idee guida condivise è una maggioranza - ne siete consapevoli anche voi - nata già morta. Per fortuna degli italiani

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, anche in occasione della presentazione del Documento di programmazione economico-finanziaria il centro-sinistra non si è smentito, esordendo con una frase di battuta da avanspettacolo, da spettacolo di intrattenimento. È stato detto infatti che quel documento, definito un manifesto economico di legislatura, può riassumersi in questo *spot*: «La scossa in tre mosse per il Paese: crescita, risanamento ed equità». Ciò rappresenta, ancora una volta,

Dopo la stagnazione dell'attività economica registrata nel quarto trimestre e nell'intero 2005, i dati relativi al primo trimestre 2006 hanno mostrato una netta ripresa.

d'improvviso, così come sono spariti gli articoli malevoli e velenosi della stampa estera, con in testa il "Financial Times", che ci accusava continuamente di una politica dissennata. Evidentemente tale politica non era dissennata, ma era una politica giusta, tant'è che il centro-sinistra, in un rigurgito di sincerità, ce ne ha dato atto e questo non può che farci piacere.

quali si dice: «Al suo interno, gli acquisti di beni e servizi scontano i contratti di fornitura (aggiuntivi al «programma Eurofighter») già stipulati dalla Difesa e derivanti anche da accordi internazionali per un impatto medio annuo superiore allo 0,1 per

al Documento di programmazione economico-finanziaria, con una maggioranza abbastanza significativa. Indubbiamente questo passaggio sul comparto della difesa non può che non solo per l'assoluta disattenzione che è stata dedicata alle problematiche del settore, ma anche per gli effetti negativi che su di esso si ritorcono.

(quelle dei farmacisti, dei tassisti, dei notai, degli avvocati, svilendo addirittura quella nobile professione) e nascondendo invece quanto vi era all'interno: mi riferisco in modo particolare alla schedatura, alla stangata fiscale, a quant'altro è stato inserito

proprio il settore della Difesa si vede impegnato su più fronti, in più campi, per il rispetto di quelle alleanze alle quali siamo legati per scelte antiche, per convinzioni democratiche, per naturale civiltà e per naturali comportamenti che abbiamo sempre tenuto e che segnano anche una continuità

demotivazione che si offre ad un comparto, quello della Difesa, ai soldati, a tutte le Forze armate, che sappiamo benissimo quanto siano impegnate e quali compiti le aspettino in un immediato futuro, specialmente dopo l'apertura degli scenari tragici del Libano. Libano. Anche su questo, dunque, vi è stato un taglio furioso, senza alcuna giustificazione; con un tratto di penna si è ulteriormente aggravata una situazione che già bella non era e che abbisognava di un miglioramento, di un segnale di discontinuità, qui sì, non rispetto al passato, dove pure erano stati fatti sforzi enormi

il Documento che stiamo discutendo oggi è sensibile ai problemi sempre nuovi dell'equità sociale propri delle società postindustriali, indica strade nuove per il *welfare* familiare, per chi è in condizioni disagiate, per gli anziani non autosufficienti e per l'infanzia. E, soprattutto, esso è sensibile al fatto che un *welfare* diverso può costituire un supporto importante della crescita e per la modernizzazione del Paese. Per esempio, un sistema di *welfare* esteso ai giovani con lavori atipici ne diminuisce la vulnerabilità, la dipendenza dalla famiglia ed accelera la loro transizione alla piena autonomia. Un *welfare* familiare che non escluda, come oggi avviene, un'importante parte della popolazione, così come una più densa ed estesa rete di servizi per l'infanzia ed un piano integrato per gli anziani non autosufficienti, è essenziale se si vuole accelerare l'accesso al mercato del lavoro delle tante donne che oggi ne stanno fuori o al margine, accesso essenziale per ricondurre il Paese su un sentiero stabile di crescita. Eppure anche questo non basterà, come si può evincere indirettamente dalle cifre contenute nel DPEF, sulle cui implicazioni vorrei attirare l'attenzione dei colleghi e del Governo. La pur moderata crescita del PIL prevista implica un aumento sia dell'occupazione, sia della produttività. Della prima si stima l'aumento in circa 700.000 unità nel quinquennio, della seconda un ritorno ad una crescita annua dello 0,7 obiettivi sicuramente ragionevoli. Ebbene, nel prossimo quinquennio la popolazione in età attiva del Paese, tra i 20 ed i 65 anni, in assenza di immigrazione diminuirebbe di circa 800.000 unità; nella componente più giovane, tra i 20 ed i 45 anni, la diminuzione sarebbe addirittura pari a 1.800.000 unità. E' vero che giovani, donne ed anziani fuori del mercato del lavoro costituiscono un serbatoio potenziale di risorse umane, ma i dati dimostrano che esso ha una limitata capienza, e l'esperienza suggerisce che ad esso si può attingere solo con gradualità. Solo una consistente e ulteriore immigrazione, numericamente equivalente a quella di anni recenti dell'ordine di 300.000 unità all'anno, può permettere all'economia di mantenere il moderato passo previsto. Qualora, nel quinquennio o successivamente, l'economia accelerasse il passo, anche la domanda di lavoro immigrato gli terrebbe dietro. I servizi alla persona, le costruzioni, il turismo, e tante altre attività ad alta intensità di lavoro sono i grandi richiedenti del lavoro immigrato; come si sa, molti settori prosperano nuotando nel sommerso, attraendo manodopera irregolare e, per sua natura, flessibile al massimo. una società con un *welfare* poco generoso per le famiglie, come quello italiano, dove la cura dei bambini, dei non autosufficienti e dei molto anziani è in gran parte delegata alla famiglia, domanda quantità crescenti di lavoro per aiuto domestico, soprattutto se questo è a basso costo. Il forte, e forse crescente, afflusso di immigrati induce ad elaborare una politica diretta a sostenere azioni incisive di integrazione-interazione, di riqualificazione e formazione, di sostegno alla mobilità sociale delle prime e delle seconde generazioni di immigrati. Sappiamo che i Paesi meno ricchi e quelli poveri che gravitano nell'orbita europea hanno potenzialità quasi inesauribili di fornire lavoro, almeno per qualche decennio, per alimentare senza problemi la nostra economia, con lavori generalmente collocati nelle fasce più basse e con deboli prospettive di promozione sociale, fattore non ultimo della deludente *performance* della produttività del sistema negli ultimi anni. E' su questo tema che occorre riflettere per mettere a punto le giuste politiche, che tra l'altro valorizzino la risorsa immigrazione senza relegarla nei settori a più bassa produttività. politiche che possono esplicare i loro effetti solo nel lungo periodo, e che potremmo collocare in varie direzioni. La prima di esse riguarda la riforma incisiva e moderna del *welfare*; le strutture per l'infanzia, la scuola a tempo pieno, i servizi integrati per gli anziani possono moderare e riqualificare la domanda di lavoro domestico e per i servizi alle persone: in breve, meno badanti e più personale specializzato. Per quanto concerne la seconda: una politica vigorosa di prosciugamento del sommerso, che tagli le gambe all'immigrazione irregolare, quasi sempre impiegata in mansioni di basso livello. Più forte e diffuso è il sommerso, più alta è la quota di irregolari tra gli immigrati: una quota che è bassa nel Nord Europa e alta nei Paesi euromediterranei. La terza politica prevede un sostegno ai processi di modernizzazione delle attività produttive, volto ad accrescere attività produttive, volto ad accrescere la produttività e che ha come effetto un alleggerimento della quota della domanda di lavoro poco qualificato. Infine, le politiche migratorie dovranno porsi il problema di come incentivare l'immigrazione con alte qualifiche, oggi fortemente scoraggiata dalle regole vigenti, e di qualificare, o riqualificare, le prerogative e capacità degli immigrati di prima generazione, sostenendo altresì i processi formativi delle seconde generazioni.

rispetto al Governo di centro-destra. Si parla di crescita, di risanamento dei conti e di equità sociale e territoriale oltre che di un quadro realistico e preoccupato dei conti pubblici. E' opportuno cominciare a declinare queste parole e questi obiettivi per indicare la strada, o le strade, all'interno delle quali il Governo dovrà muoversi con la prossima legge finanziaria anche per superare, o affrontare, con pacatezza le ambiguità che rischiano di compromettere la valenza positiva del documento alla nostra attenzione. Voglio affrontare nel merito alcuni nodi rilevanti. Il primo il concetto, ribadito più volte, della crescita e della competitività del Paese. E' un tema rilevantissimo e positivo, che non può ridursi alla promozione di uno sviluppo insostenibile,

Il Documento parla apertamente di provvedimenti che non dovranno impoverire le azioni di solidarietà, di promozione della crescita, di fornitura ai cittadini di beni pubblici essenziali. Parole opportune, che non ci rassicurano pienamente anche se comprendiamo che non si può, e non si deve, semplicemente difendere l'esistente e le sue inefficienze ma si devono trovare strade innovative per affrontare i problemi nuovi e vecchi che ci vengono posti. Voglio fare un esempio: sempre più insistentemente si parla di innalzamento dell'età pensionabile per le donne senza riconoscere in questo confronto il carico supplementare di lavoro, quantificato anche dalle statistiche, che le donne sostengono. Una proposta formulata in modo così freddo è veramente inaccettabile. Se si propone, e lo si fa soprattutto nei confronti delle donne, di utilizzare in modo più flessibile il rapporto tra tempo di vita e tempo di lavoro secondo le esigenze personali e di carico familiare;

che riconoscere nuovi problemi e dare nuove opportunità ai cittadini e alle cittadine del nostro Paese con una forte concertazione con le parti sociali sia l'unica strada per fare passi avanti e per non alimentare solo inutili conflitti nel Paese. terzo ed ultimo argomento sul quale voglio soffermarmi è il tema delle infrastrutture. E' vero, ed è già stato sottolineato, che nel Governo esistono accenti diversi sul tema delle infrastrutture.

debito pubblico anche futuro. Quindi - ripeto - c'è una forte discontinuità che desidero evidenziare. Si parla di uso efficiente delle risorse pubbliche, della necessità di selezionare la lunga lista degli investimenti, di procedure ordinarie per la TAV in Val Susa, di rivedere le regole in materia di concessioni autostradali. Si tratta di positivi ed utili segnali e di passi in avanti

diversi che vi sono in tema di infrastrutture. C'è un confronto molto aperto, ma ci sono anche linee di indirizzo molto chiare sia in questo Documento che nel programma dell'Unione con cui ci si è candidati a governare il Paese. Chiediamo di parlare di più di mobilità sostenibile e di coerenza tra politica dei trasporti ed infrastrutture. In tal senso un ruolo primario dovrà giocarlo il Ministro dei trasporti che ha annunciato un aggiornamento del piano generale dei trasporti e della logistica. di mettere le città - troppo debolmente riproposte in questo Documento - e la mobilità urbana al centro dell'agenda politica del Governo. Quelle città dove vivono e si spostano milioni di cittadini ogni giorno, con grandi difficoltà.

senza dimenticare che anche al Nord vi sono problemi seri di mobilità, di servizi al cittadino, di trasporto per i pendolari che hanno bisogno di regole, di incentivi, di processi di liberalizzazione, e anche di risorse.

Stiamo parlando di provvedimenti e di misure concrete e praticabili che sono l'asse costitutivo del programma di Governo dell'Unione. In sostanza, un modo diverso per aumentare la fiducia e rispettare gli impegni tra cittadini e politica

Signor Presidente, onorevoli colleghi,

Per quanto riguarda il contesto economico, le proiezioni del Ministero dell'economia e delle finanze segnalano che gli indicatori, che anticipano il ciclo economico mondiale, sono tutti positivi ed evidenziano una crescita costante. Questa crescita risulta più accentuata negli Stati Uniti e nell'area asiatica, mentre esiste ancora un ampio divario tra la crescita italiana e quella degli altri Paesi dell'area dell'euro. In tale contesto anche la fiducia delle imprese e delle famiglie risulta positiva; questo è chiaramente un altro segnale incoraggiante per il rilancio dell'economia. In questa fase congiunturale favorevole occorre sostenere la domanda interna (che si trova già su livelli positivi), mentre è necessario rilanciare il rapporto commerciale con l'estero, attualmente negativo. Questo *trend* negativo in realtà, più che da una fase congiunturale, dipende da una profonda crisi del sistema produttivo italiano; crisi più accentuata nell'ambito di quei settori che sono maggiormente esposti alla concorrenza internazionale. In sostanza, gioca a sfavore del sistema produttivo italiano un costo unitario per prodotto ancora troppo alto rispetto ai mercati internazionali. Quindi, Quindi, per sostenere il sistema produttivo è necessario intervenire sui fattori strutturali che determinano il costo economico dei nostri prodotti: costo del lavoro, costo dell'energia, eccessiva burocrazia, costo ed efficienza dei servizi, ritardo infrastrutturale. Dicevamo che è necessario mantenere questo clima di fiducia sia nelle famiglie sia nelle imprese. La nostra preoccupazione però è che l'azione del Governo in realtà possa scalfire questo sentimento, determinando una contrazione dei consumi e degli investimenti. Le misure adottate da Visco e da Bersani comportano inevitabilmente un aumento della pressione fiscale, mascherato da lotta all'evasione. Potrebbero addirittura far pensare ad un Grande fratello fiscale, evocato ad esempio dall'obbligo per le banche di comunicare all'Agenzia delle entrate tutti i movimenti superiori a 1.500 euro. Questo clima di percepibile oppressione fiscale, insieme alle onerose formalità burocratiche cui saranno sottoposte tutte le attività produttive, potrebbe determinare un sensibile aumento dei costi ed una perdita di competitività, soprattutto degli artigiani, delle piccole e medie imprese, dei commercianti: il vero cuore del sistema produttivo italiano. Inoltre l'aumento generalizzato della tassazione sugli utili da capitale e sugli immobili, quello ipotizzato dell'IVA, e il ritorno della tassa di successione comporteranno un effetto negativo ed una presumibile fuga di capitali e di investimenti esteri. Con le misure adottate avremo certamente un aumento della tassazione diretta ed indiretta sulle famiglie, che comporterà una riduzione dei consumi e quindi una contrazione della domanda interna. Avremo inoltre sicuramente un aumento dei costi di produzione per le imprese, con ulteriore perdita della capacità di fare concorrenza e conseguente diminuzione delle esportazioni, giacché l'intervento sul cuneo fiscale potrebbe essere sicuramente una risposta a questo problema, ma la vacuità della proposta e le sue possibili declinazioni non ci convincono, perché comunque la sua copertura finanziaria incide in modo depressivo sul quadro dell'economia nazionale, creando più problemi di quanti ne risolva. Insomma siamo in presenza di una serie di misure, adottate o annunciate, che vanno ad incidere negativamente su quel clima di fiducia esistente e necessario per rilanciare appieno il motore economico. D'altronde il decreto-legge n. 223 del 2006 contiene misure tese per i quattro quinti alla realizzazione di maggiori entrate e, per solo un quinto, alla determinazione di minori spese correnti, con una correzione pari solo allo 0,1 per cento Questa è la dimostrazione della debolezza politica di questo Governo. Le forti differenze politiche tra le forze che sostengono il Governo hanno impedito allo stesso di intervenire in maniera strutturale sul problema della spesa pubblica; a questo punto è divenuto necessario appesantire il carico fiscale che grava sulle famiglie e sulle imprese. A questa soluzione ne avremmo preferito un'altra: una riduzione qualitativa della spesa pubblica, ad esempio incidendo sulla copertura finanziaria dei servizi pubblici, attraverso una seria opera attraverso una seria opera di liberalizzazione, di apertura effettiva alla concorrenza. Per questo riteniamo necessario agire sui fattori strutturali che comportano l'aumento della spesa pubblica piuttosto che andare a colpire le famiglie e le imprese, rischio di compromettere il ciclo favorevole di crescita economica. L'aumento del rapporto qualità-prezzo del servizio, la diminuzione generalizzata dei costi per servizi sostenuti dai cittadini è la strada che consente la liberazione di risorse pubbliche da impegnare, magari nel settore dei servizi sociali. Inoltre consentirebbe ai cittadini maggiori opportunità di risparmio con un aumento potenziale dei consumi e, quindi, un miglioramento del ciclo produttivo. Una seria politica di liberalizzazione nel settore dei servizi avrebbe avrebbe effetti positivi anche sul mondo delle imprese: non dimentichiamo che il costo dell'energia è tra i più alti in Europa e incide in maniera significativa sul costo finale dei prodotti *made in Italy*. Cosi come incide sulla competitività della nostra economia il ritardo nello strategico settore delle infrastrutture: ritardo che l'Italia sconta ormai da anni e che sta determinando, in particolare in alcune zone, situazioni di oggettiva insostenibilità. Anche sul tema delle infrastrutture, e certamente in maniera non secondaria, si gioca il destino della nostra economia e delle sue potenzialità di sviluppo. Anche qui si delinea una diversa visione del problema e dei conseguenti interventi da programmare. Una differenza di valutazione da tempo caratterizza i due diversi schieramenti politici. Il centro-destra ritiene che, in una congiuntura economica mondiale favorevole, il risanamento debba strutturarsi principalmente sulla crescita e non viceversa, come

A tale riguardo il ministro Di Pietro si è limitato a presentare, nell'apposito allegato infrastrutture, una tabella meramente descrittiva e divisa in due parti: nella prima viene indicato lo stato di attuazione delle opere e degli interventi previsti dalla legge obiettivo; nella seconda

Il centro-destra ha creduto con decisione nel carattere fortemente innovativo della legge obiettivo, rilanciando con questo strumento il tema delle infrastrutture, e quindi procedendo alla individuazione delle priorità nel quadro di un grande progetto nazionale di adeguamento e di potenziamento della complessiva dotazione infrastrutturale. In tale modo, non vi è stata una sottovalutazione delle problematiche finanziarie; indubbiamente c'era e c'è consapevolezza che sono state avanzate molte proposte in relazione alla disponibilità finanziaria effettiva. Ma tali proposte possono trovare nella necessaria gradualità esecutiva, oltre che temporale, degli interventi previsti, quelle adeguate risposte in termini di concreta realizzabilità alla luce delle disponibilità attuali e prevedibili in futuro. Per quanto riguarda, invece, le infrastrutture secondarie,

locali, non venga vanificato, parzialmente o totalmente. Noi riteniamo che le priorità di intervento non possano essere dettate solo dalla singola ed immediata disponibilità finanziaria, ma che sia anche necessario prendere

è quello di condannare per molto tempo, se non definitivamente, al degrado socio-economico alcune zone del Paese per le quali l'eventuale realizzazione dell'opera prevista rappresenta una necessità non ulteriormente rinviabile. A nostro avviso, proprio nell'ottica di ridare impulso allo A nostro avviso, proprio nell'ottica di ridare impulso allo sviluppo economico e produttivo, è necessario un maggiore coraggio negli investimenti, ricorrendo, per quanto consentito ed opportuno, anche ad un maggiore apporto delle risorse private attraverso gli innovativi strumenti della finanza di progetto. In conclusione, ci saremmo aspettati dal Governo delle scelte di politica economica più coraggiose e con maggiore attenzione al rapporto qualità - quantità degli interventi. Ai buoni propositi

parlamentare con l'aspettativa di trovarle nelle norme della prossima finanziaria. In ogni caso daremo comunque, come oggi, il nostro contributo di idee e soluzioni per un'opposizione costruttiva e responsabile al servizio dell'Italia.

i settori di mia competenza (scuola, università, ricerca, cultura e turismo) è pieno di buone intenzioni, come d'altro canto tutti i documenti di programmazione economico-finanziaria.

si sottolinea l'esigenza della valutazione dei risultati (ma, anche qui, la riforma della valutazione del sistema universitario è stata avviata dal ministro Moratti); si sottolinea l'importanza della competizione fra Atenei, nella logica già indicata dal precedente Governo; si auspicano si auspicano la defiscalizzazione dei contributi dei privati alle università ed ai centri di ricerca ed una maggiore internazionalizzazione.

l'altro, la riduzione da un decimo ad un diciottesimo del costo della deducibilità delle quote di ammortamento relative ai marchi di impresa per quanto riguarda la cessione del marchio, una tassazione, dunque un inasprimento fiscale complessivo sui marchi. In merito all'internazionalizzazione, d'altro canto, è curioso come, proprio nel decreto, si preveda un taglio delle borse di studio per gli studenti stranieri:

uno dei primi provvedimenti a firma del ministro Mussi prevede il blocco del decreto sulla programmazione, che implicava un riparto delle risorse alle università proprio sulla base della maggiore efficienza nell'ambito della spesa effettuata:

a pag. 35 si legge che «Le retribuzioni pubbliche sono state valutate scontando gli effetti connessi alla corresponsione dell'indennità contrattuale, ecc.». Ciò vuol dire, forse, che sino al 2011 non vi saranno rinnovi contrattuali?

Documento, fatto di buone intenzioni e contraddetto dai primi atti del Governo Prodi, è poco incoraggiante per il futuro della nostra ricerca, della nostra scuola, della nostra università e della nostra cultura.

Presidente, vengo da una manifestazione spontanea dei farmacisti romani in piazza Barberini. Si sta creando un clima di tensione ed

ci consegnano una situazione economica e sociale pesante, in cui il peggioramento dei grandi dati dell'economia si accompagna ad una sofferenza sociale diffusa, caratterizzata da un'erosione del potere di acquisto dei salari e ad un ingigantirsi delle situazioni di precarietà e di insicurezza. I ceti medi, quelli continuamente oggetto delle attenzioni verbali della minoranza, hanno subito anch'essi gli effetti dell'acuirsi delle disparità economiche, per cui solo una piccola parte ha potuto cogliere il vento buono, naturalmente per loro, delle nuove occasioni di guadagno, in gran parte speculative,

Parte da qui, scegliendo però una via inedita, quella di mettere in relazione temporale, ma anche funzionale, l'azione tesa a produrre il rilancio dell'economia con l'obiettivo di una nuova equità sociale. Un principio ed una scelta imposti, non solo da una questione di giustizia sociale, pure ineludibile, o dalla necessità di ristorare chi in questi anni ha visto messa in discussione la possibilità di mettere insieme il pranzo con la cena, costretto da un salario troppo piccolo o magari da un mese troppo lungo. lungo. Un principio ed una scelta dettati invece anche da una interpretazione della natura stessa della crisi, basata sulla riduzione dei consumi di massa e sulla crescita incontrollata della rendita finanziaria, che ha sottratto risorse all'economia reale, alla produzione di beni e di reddito da lavoro. La relazione tra rilancio ed equità è il punto chiave del programma dell'Unione. È un elemento costituente della stessa alleanza ed è per noi un punto chiave di questo Documento, su cui dovremo impegnarci a vigilare anche e soprattutto nella successiva fase attuativa. È lo strumento attraverso cui si reimmettono nel circuito dell'economia risorse umane ed economiche che sono state escluse o lasciate ai margini pur di garantire sempre più privilegi a sempre meno cittadini. Questa nostra aspirazione ci aiuta anche nella necessaria riconnessione tra la politica e la realtà. Essa rappresenta la via attraverso cui gli elementi di macroeconomia tornano a parlare della condizione materiale di donne e di uomini; consente che entrino finalmente nella nostra discussione i rumori ed i profumi delle cose reali. Sono cose reali e concrete la diminuzione del cuneo fiscale (di cui una parte a vantaggio dei lavoratori), l'impegno per la restituzione del *fiscal* *drag*, l'impegno ad incentivare lastabilizzazione del lavoro, un rilancio delle politiche abitative, l'introduzione del reddito minimo di ingresso e l'impegno al recupero di risorse finalmente attraverso l'attacco all'elusione e all'evasione fiscale. Ieri sera, signor Presidente, è stata esposta su un banco di quest'Aula una treccia d'aglio, non destinata - almeno credo - ad una improbabile ed estemporanea bagna cauda; ritengo piuttosto volesse significare la volontà di esorcizzare l'avvento di un nuovo "Dracula fiscale". Nonabbiano timori i giovani precari, i lavoratori dipendenti, i piccoli commercianti ed artigiani: sono già stati dissanguati dalla crisi economica in cui è stato gettato il Paese; hanno semmai da meritarsi e da aspettare una trasfusione, che paghi finalmente chi non ha mai pagato. Tale obiettivo non è solo di quella parte che ha scelto di dare il proprio consenso all'Unione, ma accomuna anche molti cittadini che hanno scelto la vostra parte, colleghi della minoranza, esclusa naturalmente quella quota non piccola ma certo minoritaria che vi ha sostenuto proprio nella speranza che si continuasse a garantire il sistema dell'impunità e dei condoni. Ancora, sono cose concrete e reali, sebbene immateriali, la valorizzazione della ricerca, della scuola e dell'università, l'impegno verso uno sviluppo rispettoso dell'uomo e dell'ambiente, l'equità come risorsa per l'economia, l'equità tra i sessi, tra le generazioni, tra le classi sociali, ma anche tra i territori, quelli più fortunati e quelli più svantaggiati; prima di tutto, vi è l'attenzione al Sud, al nostro Mezzogiorno, al tentativo di riattivare i grandi giacimenti culturali, ambientali ed umani, soffocati dall'incuria e spesso dall'egoismo regionalistico miope ed inefficace.

che ha contraddistinto il rapporto tra i Gruppi della maggioranza; si è trattato di una relazione dialettica tra conflitto e compromesso che è riuscita a licenziare un Documento che nessuno può rivendicare come totalmente proprio, ma che nessuno può sentire come estraneo, che sta - appunto - su un terreno comune che ci siamo conquistati a partire dal confronto sulla proposta programmatica dell'Unione. Si tratta di un terreno che Rifondazione Comunista, pure

vi ringraziamo per aver dato atto, con il vostro Documento di programmazione economico-finanziaria relativo che l'andamento della crescita, limitatamente al periodo 2006-2007, merita di essere considerato buono; non così la previsione per gli anni successivi 2008-2011. Ciò evidentemente dovrebbe far riflettere il Parlamento, e per quanto ci riguarda il Senato, sul perché, perlomeno per l'immediato futuro e per il tempo che va, le cose si sono esternalizzate con un andamento favorevole dell'economia. Se ciò è accaduto, evidentemente non è ascrivibile ai provvedimenti che sono stati adottati all'inizio di questa legislatura e che avete intenzione di adottare, ma è ascrivibile certamente alle politiche economico-finanziarie del Governo che ha retto questo Paese nel passato quinquennio. E allora, ecco, il dubbio dovrebbe assalirvi, amici del Governo, in una logica che deve vedere certamente anteposto l'interesse generale all'interesse di partito e di coalizione. Quali sono i motivi per cui questo risultato favorevole, che oggi cogliamo per effetto di provvedimenti precedenti, si è verificato? Abbiamo capito che dall'inventario che avete fatto con questo Documento vi siete resi conto che ricorre la necessità di ridurre la pressione fiscale, di incrementare la spesa per investimenti, di contenere la spesa corrente. È una sorta di regola, o di insieme di regole, che ha fatto perdere il sonno a chi ha governato questo Paese in passato. Qualcuno ha tentato di affrontare l'argomento inerente la riduzione della pressione fiscale e lo ha fatto preliminarmente riducendo la spesa corrente, ma chiamando a governare questo processo anche gli enti locali. Con le ultime norme con le quali abbiamo stabilito che la spesa poteva essere dilatata nella misura del 2 per cento circa abbiamo chiesto il coinvolgimento e la corresponsabilità degli enti locali, di quell'esercito di amministratori che sono impegnati in prima linea sulla trincea del rapporto con l'utenza e con la cittadinanza italiana di giorno in giorno. Quindi, non ci arrogammo il diritto di contenere *tout court* con tagli che evidentemente voi volete riprendere come regola e abitudine ordinaria, ma dicemmo a quegli amministratori: governate la spesa, però sappiate che c'è un *budget* al di là del quale non possiamo andare. Voi ritenete di poter ridurre la pressione fiscale con la lotta all'evasione e all'elusione. Noi riteniamo che quel che si poteva fare anche con il Governo precedente è stato fatto e vi diciamo: non vi illudete che per quella via riusciate a trovare tante risorse senza deprimere il sistema produttivo, che già di per sé è depresso e per la cui rivitalizzazione lavorammo non poco. Lungi da noi il pensare che non bisogna fare la lotta all'evasione, ma non ci possiamo illudere che ammazzando il malato si migliori la qualità della vita del popolo italiano sotto il profilo fiscale.

si dovette verificare che questo Paese non aveva più propensione all'esercizio dell'attività di impresa e di lavoro autonomo. Se ciò dovesse accadervi certamente quella crescita che avete inventariato per il 2006-2007 non ci sarà più per il 2008-2011. Vi diciamo con la logica e l'impegno di chi quanto voi è parlamentare e certamente non vuole vaticinare insuccessi ma solo esprimere le sue preoccupazioni: state attenti, perché vi potreste di nuovo ritrovare con un sistema produttivo che ha bisogno della rianimazione, così come fu quello che ci consegnaste nel 2001. Con riferimento alla spesa per investimenti in questo Paese è storica la pratica di rivitalizzare il sistema con la spesa pubblica. La spesa pubblica per investimento era la terapia che abbiamo praticato e che vi ha dato anche un buon risultato di crescita per il 2006-2007. State attenti

pugliese, quella del Ponte sullo Stretto non diviene una spesa o un progetto da considerare fuori luogo e fuori dai tempi ma quanto ci vuole per la circuitazione di uomini e mezzi nel Mezzogiorno d'Italia, d'Italia, quel Mezzogiorno del quale avete detto che volete migliorare la condizione di vita. Tutto è possibile, ma rimangono e rimarranno desideri se non ascolterete e guarderete la storia economica, che è maestra di vita, non perché fatta da noi nell'ultimo quinquennio, ma perché senza la lettura della storia economica non si può costruire un buon avvenire. Tanti auguri. Ci auguriamo che le cose non vi vadano così male, ma non per voi, quanto per il popolo italiano, del quale evidentemente tutti siamo espressione.

Il Documento in esame propone alla nostra attenzione, infatti, il dato di una ripresa congiunturale nel corrente anno. Senza dubbio una situazione positiva, pur in presenza di un quadro europeo che manifesta stime di crescita superiori alle nostre. In ogni caso, la ripresa congiunturale è evidenziata dal fatto che la stima del tasso di crescita del prodotto interno lordo, pari all'1,5 per cento, è persino superiore al tasso di crescita potenziale della nostra economia, fissato a circa l'1,2 Questi dati offrono quindi un quadro caratterizzato da una possibile ripartenza della nostra economia dopo anni nei quali lo «zero virgola» ha segnato il tasso di crescita del Paese. D'altra parte, però, va assunto con particolare attenzione il quadro complessivo della finanza pubblica attestata in un perdurante stato di gravità, come evidenziato dal livello dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione, pari a quasi il 4 per cento nel 2006, pur in presenza di un possibile impatto favorevole determinato dalle stesse misure previste nel decreto-legge n. 223 che ieri è stato approvato La situazione dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione non può non preoccupare, tanto più in considerazione del fatto che, nell'ipotesi confermata di un tasso di crescita dell'economia italiana pari all'1,2 per cento nel periodo 2007-2011, tale indebitamento netto è destinato a rimanere costante nel tempo se non saranno attuati decisivi e strutturali interventi su questo delicatissimo fronte. sicuramente allarmante; le previsioni in questione si basano infatti sulla legislazione vigente, sottostimando così l'andamento della spesa pubblica poiché non si possono al momento considerare, ad esempio, gli incrementi derivanti dagli oneri contrattuali del personale. Diventa perciò certamente ineludibile la messa in campo di interventi strutturali che mirino a ridurre, o perlomeno a comprimere, il livello di spesa pubblica con particolare riferimento a quella corrente. Si tratta, quindi, di operare con convinzione verso la ricostituzione di un avanzo primario permanente e da qui anche la consapevolezza di necessari interventi di natura strutturale. Risulta quindi a mio parere opportuna la scelta di adottare stime di crescita del prodotto intorno lordo prudenti e realistiche. Ciò consente, soprattutto sul versante delle entrate, di evitare previsioni troppo o forzatamente ottimistiche che potrebbero risultare non sempre facilmente realizzabili. Del Documento è quindi importante e doveroso richiamare l'innovazione culturale e politica dettata dall'individuazione di linee strategiche che abbracciano l'intera durata della legislatura chiamando così tutti, in particolare Governo e Parlamento, ad una maggiore e più trasparente assunzione di responsabilità politica. Risulta perciò importante e sicuramente meritevole di segnalazione in questo dibattito il dispiegarsi della strategia di politica economica della maggioranza per gli anni 2007-2011 sul triplice fronte, appunto, della crescita, del risanamento e dell'equità, come ieri ha ricordato lo stesso ministro Bersani nel suo intervento di replica nel dibattito sulla conversione in legge del decreto-legge n. 223. In ogni caso, si tratta di un vero proprio fronte unico, articolato su tre linee di intervento strettamente correlate tra loro, su cui investire complessivamente ogni impegno per il rilancio generale del nostro Paese. Come detto in precedenza, quindi, risulta fondamentale e condivisibile - in questo contesto - la scelta di privilegiare interventi strutturali, per ricostruire un avanzo primario permanente, così come va evidenziato l'obiettivo e il conseguente impegno a ridefinire le regole che attengono al rispetto del Patto di stabilità interno. A tale proposito, credo vada fatta osservare la proposta di tornare ai vincoli sui saldi, anziché sui limiti basati sui tetti di spesa. A monte di questa proposta vi è l'assunzione, certo tutta politica, ma direi anche culturale, di aprire una fase nuova nell'obiettivo di valorizzare e tutelare l'autonomia finanziaria degli enti territoriali. In questo contesto, si palesa, e si rende perciò evidente, il progetto teso a rendere effettivi e praticabili gli strumenti del federalismo fiscale, chiamando in ogni caso tutti i livelli istituzionali ad un rapporto trasparente e di reciproca responsabilità. Il Documento di programmazione economico-finanziaria presenta un ulteriore significativo punto programmatico. È un punto di grande importanza, dettato dalla scelta di prevedere una riduzione della pressione fiscale, pur in un quadro in cui si evidenzia con decisione l'obiettivo del contenimento della spesa pubblica. Il contesto in cui si manifesta questa scelta è dato dalla volontà di favorire una più equa distribuzione dell'onere fiscale. Tutto ciò attraverso precise azioni finalizzate al contrasto dell'evasione e dell'elusione. queste azioni è certamente quello di promuovere un maggior equilibrio nel prelievo, secondo le diverse tipologie di reddito. È una scelta essenziale per ristabilire nel nostro Paese condizioni di effettiva equità ed equilibrio sociale

Presidente, il DPEF disegna il quadro generale degli interventi da attuare attraverso la successiva manovra finanziaria e di bilancio. È necessario quindi aspettare e verificare la traduzione delle linee presenti in questo Documento in impegni concreti nella legge finanziaria. Documento al nostro esame ci sono luci ed ombre, per usare un'immagine pittorica: di queste luci ed ombre desidero affrontare alcuni argomenti che mi sembrano importanti. importanti. In coerenza con il programma dell'Unione, la politica economica deve essere orientata a perseguire contemporaneamente i tre obiettivi del risanamento, dello sviluppo e dell'equità sociale e territoriale, perché i nostri elettori ed elettrici, lavoratori uomini e donne, precari ed intermittenti, pensionati e migranti hanno in questo ultimo ventennio già pagato un alto prezzo in termini di dignità e sicurezza della loro condizione e non possono essere chiamati ad altri sacrifici. Per quanto concerne l'aspetto del risanamento dei conti pubblici, auspichiamo e ribadiamo che il percorso di rientro del *deficit* sia modulato in tempi tali da contenere e ridurre il più possibile eventuali tagli alla spesa sociale ed agli enti locali - che degli interventi sociali sono i primi attori mentre bisogna far leva sulle entrate con la lotta all'evasione e all'elusione fiscale e contributiva, operando, lo sottolineo, più sulle entrate che sui tagli. Per questo sono necessari interventi mirati ad uniformare la tassazione sulla rendita finanziaria, sui grandi patrimoni e ripristinare il principio della progressività dell'imposizione diretta così come previsto dalla nostra Costituzione, Se di tagli dobbiamo parlare, vorremmo che questi riguardassero piuttosto le spese militari con una politica di disarmo e di riduzione delle spese militari stesse, bloccando le costruzioni di nuovi sistemi d'arma, rivisitando il finanziamento alle missioni militari, sostenendo la riconversione dell'industria bellica e finanziando in misura sufficiente il servizio civile nazionale, importante occasione esperienziale per ragazze e ragazzi. Per quanto riguarda gli interventi per lo sviluppo economico e la crescita, questi devono essere coniugati e non possono prescindere dalla valutazione della loro sostenibilità ambientale: sotto questo aspetto, significativa e positiva è l'introduzione di indicatori ambientali a fianco dei tradizionali indicatori macroeconomici, l'introduzione di un sistema di compatibilità ambientale e l'impiego della Valutazione ambientale

Per inciso, la medesima valutazione sull'impatto sociale delle politiche è da adottare sui temi della povertà e dell'istruzione, ma anche sull'inclusione delle categorie svantaggiate, l'immigrazione, i diritti fondamentali, l'accessibilità ai servizi e le pari opportunità. Tornando al tema dello sviluppo economico e dell'ambiente, nel DPEF si fa riferimento all'applicazione del Protocollo di Kyoto, anche se devono essere evidenziati gli strumenti operativi. Tra questi, è da sottolineare l'urgenza di introdurre il Piano energetico nazionale, fondamentale per il suo intreccio con lo sviluppo industriale; altresì importante è la Conferenza sull'energia. Nel Documento si afferma che il rilancio dell'economia passa attraverso l'aumento della produttività e del lavoro: una delle questioni per noi centrali è il superamento, non la rivisitazione, come dice il Documento, della legge n. non solo nell'abrogazione di alcune tipologie di lavoro come il lavoro a chiamata o lo *staff leasing*, forme eclatanti, estreme e tra le meno utilizzate, ma in una azione di contrasto della precarizzazione del lavoro diretta a ridurre anche l'impiego di co.co.pro. e le cosiddette partite IVA e quindi a promuovere forme di lavoro stabili, a tempo indeterminato, e a contrastare il lavoro nero e irregolare. È evidente, per quel che riguarda il lavoro sommerso, che leggi che consentano linearmente e semplicemente la regolarizzazione ai cittadini migranti, come il permesso di soggiorno per ricerca di lavoro e lo *sponsor*, per esempio, sono decisive per l'emersione del lavoro sommerso, oltre che per riconoscere dignità di cittadine e cittadini a questi produttori di ricchezza e di benessere e sottrarli alla estrema ricattabilità cui li condanna l'irregolarità amministrativa. Determinante sarà anche la valorizzazione del lavoro di cura, in particolare femminile, svolto da quelle che sono state definite badanti e che oggi molto correttamente si propone di rinominare assistenti domiciliari attraverso il miglioramento delle condizioni contrattuali, della formazione e della qualificazione professionale. Per quanto concerne le politiche per l'equità e la giustizia sociale, queste non devono essere confinate al solo contrasto dell'emarginazione, della fragilità e della vulnerabilità sociale, pur necessario ed urgente e per il quale bisogna garantire un aumento del Fondo sociale e delle risorse consegnate agli enti locali per lo sviluppo delle pratiche di contrasto alla povertà, ma devono riguardare anche misure volte all'occupazione e direttamente redistributive, mirate ad elevare le condizioni di vita di lavoratori e lavoratrici, pensionati e disoccupati. Non moderazione salariale, ma aumento del potere d'acquisto di stipendi e salari, invertendo quella tendenza ventennale alla diminuzione continua dei redditi che ha portato alla prostrazione di larghi strati della popolazione. Quindi, bene, benissimo gli interventi di conciliazione tra vita personale e lavorativa. Un consiglio: non bisogna parlare di conciliazione per le responsabilità femminili, perché altrimenti questo riconsegna ogni intervento di conciliazione al fatto che alle donne sia destinata comunque tutta la fatica, e a volte anche il piacere, dei lavori di cura. Quindi, tempo di vita e tempo di lavoro. Bene le misure di sostegno del reddito, bene l'impegno allo sviluppo della rete di servizi per l'infanzia, *in primis* gli asili nido

restituzione del *fiscal drag*, riduzione del cuneo fiscale sia per il datore di lavoro, sia per i lavoratori e le lavoratrici, senza agire sulle aliquote pensionistiche, riduzione selettiva per favorire il lavoro a tempo indeterminato, mentre sul fronte della spesa sanitaria, inferiore in Italia ancora oggi alla media europea, occorre puntare ad una stabilizzazione della spesa e non alla sua riduzione, con interventi di riqualificazione e razionalizzazione, confermando il nostro sistema di accesso universalistico alle prestazioni. quindi, che dovranno essere precisate, illuminate, con la legge finanziaria che il Gruppo di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea guarderà con grande attenzione.

facendo riferimento ad un'intervista radiofonica del ministro Padoa-Schioppa, riportava la sua preoccupazione - dice lo stesso Ministro

Lo dico non per spirito polemico, ma per cercare di argomentare rispetto ad un tema che è stato centrale nel dibattito politico elettorale che ha caratterizzato la contrapposizione tra gli schieramenti negli ultimi cinque anni almeno.

relativo allo sviluppo e alla competitività del Mezzogiorno e alla politica regionale per trovare alcune affermazioni importanti sull'azione del Governo; non di questo, ma di quello che lo ha preceduto. Si afferma che, tra la fine del 2005 e la prima metà del 2006, alcuni segnali positivi per il Sud provengono dal miglioramento dell'occupazione, dal clima di fiducia delle imprese e dal buon andamento delle esportazioni. Si cita peraltro un riferimento importante quando, a proposito della riflessione ulteriore sull'occupazione e sulla criticità del tasso di occupazione, si afferma che complessivamente i risultati raggiunti negli ultimi anni nel Mezzogiorno sono significativi, ma senza dubbio insufficienti, come è peraltro nella consapevolezza Inoltre, nel DPEF si fa riferimento ad alcune criticità strutturali, ad iniziare dalla questione della scuola, e tuttavia si riconosce e si dichiara testualmente: «nonostante i progressi conseguiti in tema di minore dispersione scolastica». scolastica». Nel DPEF si indica l'esigenza di individuare misure che determinino meno trasferimenti alle imprese e più investimenti pubblici: ciò è esattamente in linea con quanto accaduto negli ultimi cinque anni,

bisogna mantenere il livello di risorse finanziarie allo 0,6 per cento del PIL, in linea con le leggi finanziarie degli ultimi anni.

senza dare vita a quel riassetto, anche di carattere istituzionale, che meglio avrebbe consentito di governare il processo delle politiche verso il Mezzogiorno. Le altre questioni riguardano, in primo

pone continuamente il tema della cosiddetta fiscalità di vantaggio (che meglio dovrebbe essere definita fiscalità compensativa per il Mezzogiorno)

stessa centralità che nella manovra annunciata assume la questione della diminuzione del cuneo fiscale determina sostanzialmente che si tratta di una manovra che, al di là del merito,

è dimensionalmente e inevitabilmente concentrata sulla grande impresa, non certo sulla piccola o media impresa. Quindi si tratta di una manovra che non dà respiro alla possibilità

a cosa scrive oggi Pier Carlo Padoan a proposito di questa manovra e proprio per il fatto che si tratta di una misura

che ci sia una sorta di strano intreccio tra un dibattito politico piatto all'interno delle Aule parlamentari, in particolare nel centro‑sinistra, e l'enfatizzazione di alcuni temi, come è accaduto nel corso del

«non abbiamo bisogno di una ulteriore proliferazione imprenditoriale, perché essa è già iscritta nel codice genetico del nostro modello di sviluppo; abbiamo bisogno di avere qualche *big player* sul mercato dei fattori sistematicamente strategici». le piccole imprese sono fortemente competitive nel mercato, ma deboli sul mercato dei fattori e quindi avrebbero bisogno di grandi scelte strategiche su alcuni costi, ad iniziare dal tema dell'energia, e di costruire per questa via

contrasta il tessuto produttivo fondamentale di questo Paese, l'alleanza sociale maggioritaria al suo interno, per privilegiare, come sempre ha fatto il centro-sinistra, la vecchia triangolazione del potere risalente agli anni Settanta, che si esprime oggi in forme moderne in quel paradossale, ma comprensibile, blocco sociale centrato non sull'economia reale, ma sull'economia finanziaria.

è in realtà un libro dei sogni che, allo stato attuale, sembra di difficile, per non dire impossibile, realizzazione, come peraltro ha segnalato anche la relazione della Corte dei conti. Indubbiamente la promessa più ardua è quella di ricondurre il rapporto *deficit-* PIL all'interno della forbice del 3 per cento già nel 2007, con tagli su quattro grandi direttrici: pensioni, sanità, pubblica amministrazione ed enti locali. Tutto questo rispetto all'impegno della manovra che, come è ovvio, ammonta a 35 miliardi di euro, di cui 20 di minori spese e 15 di investimenti.

Credo che la declinazione di 20 miliardi di euro di risparmi e l'obiettivo strategico indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2007- 2011 di ottenere tutto questo attraverso un assunto che prevede di declinare una maggior crescita, un risanamento e un'equità siano un compito molto arduo che mi permetto di definire un libro dei sogni. Entrando nel merito di una materia che ho seguito specificatamente, chiedo, a fronte di queste premesse, dove trovare le risorse per finanziare il Fondo sanitario nazionale.

Per quanto riguarda la sanità, credo si possa evincere - d'altro canto, è anche scritto - che per recuperare le risorse non ci sono molte strade se non quella di prevedere nuove tasse, di farle imporre alle Regioni o agli enti locali, e quella di inserire *ticket* di compartecipazione. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria l'ipotesi è scritta e, di conseguenza, credo abbastanza percorribile. In modo specifico, per quelle Regioni che non lo hanno già fatto, sulla compartecipazione dei farmaci si ipotizza il *ticket* sui ricoveri. Ebbene, già paghiamo i *ticket* sui farmaci in alcune Regioni, già dobbiamo comprare i farmaci generici per risparmiare sulla spesa farmaceutica,

e credo che questo sia un po' nelle corde del Ministro - ci dirà anche di che cosa ci dobbiamo ammalare. Visto che il costo è diretto rispetto alla patologia, penso che questo Governo arriverà anche a questo In ambito sanitario - lo ricordo perché le cifre per chi ha fatto l'amministratore rappresentano un elemento di riferimento importante - le Regioni chiudono il 2006 complessivamente con un disavanzo pregresso che si accumula su varie voci (quello del 2004, quello del 2005, una compartecipazione allo sforamento della spesa farmaceutica, dove le Regioni hanno messo la loro quota e il Governo deve ancora metterla) e che si aggira all'incirca - naturalmente si tratta di dati

di 7 miliardi di euro. Se a ciò aggiungete che per il 2007 le Regioni chiedono un adeguamento del finanziamento dei LEA, le prestazioni che le Regioni si sono impegnate a fornire attraverso un accordo con il Governo ai cittadini italiani, secondo il principio, sancito dalla Costituzione, del diritto alla salute, potete immaginare che - credo e stimo

addirittura 100 miliardi di euro per finanziare il Fondo sanitario. Mi domando - pongo questo punto di riflessione - dove questi soldi dovranno essere e saranno reperiti. Aggiungete a questa cifra, stimata per far funzionare il nostro sistema sanitario, il problema, che nel vostro Documento di programmazione economico-finanziaria è comunque citato, di voler fare degli investimenti sulle nuove apparecchiature diagnostiche e tecnologie, la ripresa di una politica di investimenti sull'edilizia sanitaria, *ex* articolo 20, e naturalmente tutta la partita che riguarda l'intesa del 23 marzo 2005 per quelle Regioni che non hanno rispettato

Mi permetto di aggiungere che mi aspettavo da un Governo che fin dai primi passi ha mutuato dalla sinistra la profonda consapevolezza della propria superiorità intellettuale che la questione della sanità venisse affrontata con maggiore coraggio e lungimiranza,

alcuni dei titoli di sintesi che hanno preceduto nei giorni scorsi l'analisi fatta da molte parti sul Documento di programmazione economico-finanziaria varato dal Governo recitavano grosso modo così: le buone intenzioni ci sono, ma servono le riforme; un DPEF per arginare le disuguaglianze, un DPEF bello e impossibile; c'è rischio però che il Paese resti fermo.

concede al DPEF, nella critica dei contenuti, di aver assolutamente colto la situazione nell'analisi e di aver prospettato gli obiettivi di fondo, ma nelle tre sintesi che ho ricordato si avanza il dubbio che le azioni che dovranno essere sviluppate nel corso dell'attività che seguirà l'approvazione del DPEF nel corso della legislatura possano essere realmente realizzate. Penso che il compito del Governo e della maggioranza che lo sostiene sia quello di evitare che tale previsione di prudenza si realizzi e di accompagnare tutto ciò che seguirà al DPEF, perché gli obiettivi possano essere realizzati con le azioni conseguenti. Nell'analisi da cui si parte occorre sottolineare alcuni punti di rilievo che hanno ispirato le proposte: l'Italia nei suoi caratteristici dati di finanza pubblica è grosso modo tornata quasi dieci anni indietro. La differenza fondamentale che esiste rispetto a dieci anni fa - e non è poco, anzi direi che è il capitale più grosso che abbiamo accumulato - è che siamo dentro la moneta unica europea. Oltre a ciò, l'Italia è il Paese che, insieme al Regno Unito e agli Stati Uniti, tra i Paesi più sviluppati, condivide il primato del tasso più acuto di disuguaglianza. In altri termini, la forbice della distribuzione della ricchezza tra i più poveri e i più ricchi è tra le più elevate: il 10 per cento delle famiglie percepisce il 26,7 dei redditi prodotti al netto delle tasse, mentre il 10 per cento delle famiglie con il reddito più basso raccoglie solo il 2,6 per cento, cioè dieci volte di meno. Se si guarda al patrimonio, la distanza risulta ancora più evidente: il 10 per cento delle famiglie più ricche possiede il 43 per cento dell'intera ricchezza netta.

ed acuite nel decennio 1985-1995, guarda caso proprio negli anni in cui il debito pubblico si è sostanzialmente triplicato. Un altro elemento di analisi fondamentale che occorre tener presente e che ha ispirato sicuramente la linea del DPEF, è che le retribuzioni reali del settore manifatturiero, tra il 1995 e il 2005,

Nello stesso periodo è cresciuto a dismisura l'attivo dei redditi finanziari che, come si sa, sono in Italia sottoposti a un prelievo fiscale pari a circa la metà di quello mediamente in vigore negli altri Paesi più sviluppati, Stati Uniti compresi. L'origine di questa situazione sta in una storia travagliata che ci ha visto negli ultimi dieci anni combattere con armi diverse per stare insieme agli altri Paesi più industrializzati, usando per un periodo il tasso di cambio come leva per concorrere in aiuto alla nostra genialità e creatività - che non ci è mai mancata, anche se non è stata da sola sufficiente - e,

consapevoli che i vincoli nuovi che la globalizzazione e l'eliminazione graduale, ma costante, delle barriere di accesso ai prodotti imponeva un approccio di tipo continentale-europeo per vincere le nuove sfide che lo sviluppo ci metteva di fronte. Dobbiamo realisticamente prendere atto che siamo riusciti a fatica, finora, a stare dentro la famiglia dell'euro, ma non abbiamo contemporaneamente creato i presupposti perché la nostra economia tenesse il passo degli altri: negli ultimi cinque anni non siamo cresciuti, o siamo cresciuti troppo poco. La nostra bilancia commerciale testimonia la perdita di competitività internazionale dei nostri prodotti; prima usavamo il tasso di cambio, per difenderci, come si diceva, mentre oggi non lo possiamo più fare.

Il livello dei consumi interni, che avrebbe dovuto ricevere stimolo dalle politiche di riduzione della pressione fiscale proclamate dal Governo precedente, in realtà è rimasto stagnante, così come gli investimenti pubblici non sono stati in grado di sostenere un incremento del tasso di crescita. La disuguaglianza presente fra le aree più sviluppate e quelle in ritardo, inoltre, si è accresciuta: il Mezzogiorno continua ad essere, nello stesso tempo, il problema principale - come diciamo noi - e la fondamentale opportunità di crescita. Oggi,

Il nostro sistema economico, insieme a quello europeo, ha una sfida fondamentale da vincere con il resto del mondo industrializzato, che vede sempre più nuovi e importanti attori, in particolare in Asia: quella di produrre beni e servizi senza l'aiuto delle barriere protettive

nelle azioni da intraprendere lungo un doppio binario: da un lato concertazione di tipo istituzionale; dall'altro, concertazione con le forze sociali ed economiche che rappresentano il mondo dell'impresa, produttivo e del lavoro. L'azione si svolge, quindi, lungo tre direttrici fondamentali: proseguire, con maggiore convinzione e ulteriori azioni sulla linea della liberalizzazione e del miglioramento della concorrenza, ovviamente con occhio attento agli strumenti di regolazione, che sono fondamentali ed efficaci. Tutto questo credo possa essere realizzato - pur nelle difficoltà che registriamo anche in questa Camera - se sapremo stabilire fra maggioranza e opposizione

colleghe senatrici e colleghi senatori, molti cittadini ripongono grandi speranze nella politica economica del nuovo Governo, è alta l'aspettativa che si possano finalmente affrontare ed effettuare scelte che vadano nella direzione dell'equità e della coesione sociale. Molti cittadini italiani, anche delle classi medie e, soprattutto del Meridione, hanno sperimentato in questi anni un netto peggioramento delle proprie condizioni economiche, al punto che si parla della cosiddetta crisi della quarta settimana. Nelle aree interne del Meridione continua senza sosta lo spopolamento dei piccoli Comuni, e nuove migrazioni coinvolgono soprattutto i giovani, molti dei quali con un elevato livello di formazione, che sono costretti a trovare altrove una collocazione. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria si afferma che si deve agire simultaneamente sui tre fronti del risanamento, della promozione dello sviluppo e dell'equità; si delinea un programma che lascia intravedere la possibilità di un modello di sviluppo fondato sulla nuove tecnologie, che si relazioni in modo equilibrato con l'ambiente e il territorio, che possa portare investimenti nel sistema delle infrastrutture materiali e immateriali e anche nell'istruzione, nella formazione, nella ricerca scientifica e tecnologica. Noi speriamo che queste linee possano tradursi in una legge finanziaria che vinca la sfida di conciliare risanamento ed equità sociale; speriamo che l'esigenza di risanamento e di abbattimento del rapporto tra debito pubblico e PIL non comporti tagli indiscriminati alla spesa pubblica, in particolare alla scuola, alla sanità, al sistema pensionistico; che non comporti ulteriori dismissioni del patrimonio pubblico e ulteriori privatizzazioni. Una riduzione della spesa pubblica dovrebbe puntare sì a una maggior efficacia dell'amministrazione pubblica, ma valorizzando l'intervento pubblico e ridando senso e ruolo ai lavoratori dipendenti. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria è ribadita l'importanza che rivestono gli investimenti infrastrutturali, in particolare per il Mezzogiorno. Si afferma che è indispensabile che la spesa per gli investimenti sia riqualificata, attraverso iniziative che assicurino il rispetto di alcuni requisiti essenziali: effetti strutturali duraturi delle opere, loro attitudine a soddisfare i bisogni effettivi, certezza dei tempi di realizzazione, prevedibilità dell'impegno finanziario richiesto per l'intero arco di tempo necessario per condurle a compimento. È evidente che, come si afferma nel parere espresso dalla Commissione lavori pubblici sul DPEF, la legge obiettivo delle essere superate, oltre a una registrazione notarile e meccanica sullo stato dei progetti esistenti, bisogna individuare i criteri per fissare le priorità delle opere. Per individuare in maniera attenta i progetti infrastrutturali prioritari, è necessario un esame non solo in funzione ricognitiva ma di approfondimento delle strategie future. Le infrastrutture hanno un carattere strategico fondamentale, in particolare per il Mezzogiorno e per le aree interne. Siamo di fronte ad una qualità dei servizi del tutto insoddisfacente. Dice il Documento che la qualità dei servizi collettivi del Mezzogiorno è decisamente peggiore rispetto al Centro-Nord, dai trasporti ai settori dell'ambiente e dell'energia, dai servizi idrici all'istruzione.

la manutenzione e la messa in sicurezza della rete stradale ordinaria sono obiettivi che non possono essere elusi e che non possono essere sacrificati a favore delle grandi infrastrutture autostradali o dell'alta velocità ferroviaria. Le piccole opere sarebbero davvero grandi opere per i cittadini che quotidianamente vivono e si spostano all'interno delle nostre zone. Le risorse individuate per la realizzazione del ponte sullo Stretto, di cui dev'essere sospeso l'*iter*, potrebbero essere destinate proprio ad un piano reale di modernizzazione dei sistemi di mobilità per garantire davvero a tutti e tutte, anche ai cittadini del Mezzogiorno, anche a quelli delle aree interne, il diritto ad una mobilità di qualità. Ci auguriamo che la sfida di conciliare il risanamento, la giustizia sociale e un rilancio vero, reale del nostro Mezzogiorno possa davvero essere vinta. è a nostro avviso doveroso accompagnare la ripresa in atto proseguendo l'azione rivolta a produrre un ambiente favorevole all'impresa e alla sua attitudine a rigenerarsi in termini di maggiore competitività. Ciò significa rimuovere gli oneri impropri che gravano sul sistema produttivo italiano in termini di logistica, energia, costo del lavoro per unità di prodotto, oppressione burocratica e fiscale. Il Governo Berlusconi ha operato lungo questa linea attraverso il piano per le grandi opere, sostenuto dalla cosiddetta legge obiettivo, la diversificazione delle fonti energetiche - inclusa l'opzione del nucleare e l'impulso ad una reale liberalizzazione del mercato elettrico, le riforme per il capitale umano (la scuola, il lavoro, la previdenza, l'immigrazione), la produzione di testi unici e l'ambiziosa riforma del sistema fiscale nel segno della riduzione strutturale del prelievo e della leale collaborazione tra fìsco e contribuente. Se limiti vi sono stati, questi hanno riguardato la portata del cambiamento e, soprattutto, la sua velocità posto che, in un mercato globale così competitivo, il confronto si rivolge non al nostro passato, ma al presente dei nostri competitori. Per capirci, sarebbe stato necessario, in questo caso, un conflitto ancor più forte con la opposizione politica e sociale di allora che non ha mai condiviso alcuna delle direzioni di marcia intraprese. Ci avrebbe potuto aiutare una migliore manutenzione del Patto per l'Italia, attraverso il quale avevamo isolato le componenti più conservatrici della opposizione sociale. Ora quella opposizione si è fatta Governo e, al di là dei modi paludati del Ministro dell'economia essa già manifesta nel Documento di programmazione economico-finanziaria la sua volontà di invertire i percorsi del rinnovamento strutturale. Il polverone sul presunto squilibrio dei conti pubblici ha malamente coperto l'incapacità politica della nuova maggioranza parlamentare di proseguire molte delle grandi opere; la scelta nucleare è già negata e l'ulteriore liberalizzazione dell'energia sarà paralizzata da alcuni interessi sensibili; le riforme della scuola e del lavoro sono destinate a regredire per l'esplicita avversione alla loro implementazione e per la promessa di sostanziosi interventi correttivi; il tentativo di qualificare i flussi migratori, a partire dalla formazione-selezione nei Paesi di origine, è stato già negato dalla logica adottata della sanatoria a piè di lista degli ingressi subiti; la riforma della previdenza sarà corretta sotto il profilo della fondamentale della fondamentale previsione dell'innalzamento forzoso dell'età di pensione con conseguenze gravi per la sostenibilità del sistema pensionistico e dello stesso equilibrio di finanza pubblica; è in evidente ripresa la linea della complessità burocratica attraverso la rimessa in discussione del lavoro di semplificazione in materia ambientale e la proposizione di nuove norme, tutte segnate dalla sfiducia nei confronti della persona fisica come della persona giuridica; tutta la linea di riforma fiscale è già stata rivoltata come un calzino attraverso la negazione di ogni soluzione di leale collaborazione tra fisco e contribuente, l'affermazione di uno Stato di polizia fiscale fondato sulla delazione e su estesi poteri autoritativi dell'amministrazione senza garanzie per il contribuente, la promessa di eliminare il secondo modulo della riduzione del prelievo. Segnalo in particolare quest'ultimo profilo della politica di controriforma, non solo perché ha costituito l'intervento più corposo del nuovo Governo, enfaticamente richiamato nel lo faccio anche perché tutte le promesse di contenimento della spesa corrente sono, non a caso, indeterminate nei modi e negli effetti finanziari. Non vi è alcuna disponibilità a ripensare l'insostenibile carattere universale del Servizio sanitario nazionale; i doverosi processi di mobilità nel pubblico impiego, premessa per l'innesco di un circolo virtuoso fatto di nuovi concorsi, carriere meritocratiche, retribuzioni ancorate a risultati, sono paralizzati dal vincolo concertativo; la spesa previdenziale, per le ragioni dette, è destinata a riprendere la corsa. E in questo contesto il vero Ministro dell'economia e delle finanze sarà il vice ministro Visco, ben lieto, penso, di supplire con il maggiore prelievo fiscale all'incapacità decisionale sulla spesa. Con gli effetti ben prevedibili in termini di attitudine ad investire e competere del sistema delle imprese. Anche perché il Governo non agirà in funzione della modernizzazione del sistema di relazioni industriali, causa non secondaria della bassa produttività del lavoro in Italia. La riduzione del cuneo fiscale e contributivo, la cui copertura pare desinata a risolversi solo in termini di maggiori entrate, può costituire una leva importante per la competitività solo se sarà destinata a sostenere le componenti premiali - e quindi variabili - della retribuzione, frutto di quella negoziazione «complice» che si può sviluppare solo nel territorio e nell'impresa, lontano dalla logica della moderazione «piatta», propria della contrattazione nazionale. Si tratta di un vero e proprio rovesciamento del modello contrattuale, oggi difeso solo dalla CGIL, fondato sull'antagonismo di classe che, come tale, non determina convergenza degli interessi verso la maggiore produttività. Ma il Governo non farà nulla di ciò, prigioniero com'è delle componenti più conservatrici del sindacato e dello stesso mondo imprenditoriale. In conclusione, mi sia consentita una testimonianza sull'improprio riferimento al 1992, anno nel quale si sarebbe verificata un'emergenza della finanza pubblica analoga a quella attuale. Poiché io c'ero ed ero al fianco di Giuliano Amato in quel Governo, posso ben ricordare le straordinarie e ben diverse condizioni di allora, quando ancora c'erano la lira ed un servizio del debito pubblico particolarmente oneroso. Anche il ministro Padoa-Schioppa conosce bene quel contesto perché lo ha vissuto in un ruolo rilevante. Il fatto che egli oggi ricorra a questo improprio paragone significa solo che è già consapevole del probabile fallimento del suo Governo e, mentre i suoi colleghi Visco e Bersani si occupano degli untori cui addossare la colpa, egli cerca alibi nella lettura viziata dell'eredità ricevuta. Si tratta di comportamenti irresponsabili che impongono un'opposizione determinata a sostituire quanto prima un Governo pericoloso per il futuro del Paese.

L'elemento generale è il confronto tra il Documento di programmazione e la manovra che è stata posta in essere, perché non è possibile pensare che nel Documento sia delineata una strategia e poi non si tenga conto dei passi concreti che la maggioranza il Documento viene letto alla luce della manovra fatta, emergono tutti i limiti del Documento stesso. Con la manovra, approvata con fiducia dalla maggioranza ieri sera, il Governo ha ottenuto, tutti insieme, una serie di risultati negativi, che non sono assolutamente leggibili in maniera positiva, neppure per il futuro. Per esempio, la manovra di rientro dei conti pubblici, che è il grande impegno obiettivo del Governo, com'è noto, nel 2006 non è riuscita affatto. Non mi stanco di ripetere la manovra dei conti pubblici è cifrata dal Governo per soli 57 milioni di euro, una grandezza trascurabile, e tutto viene rinviato agli anni successivi. Vedremo allora cosa accadrà. Di certo quest'anno i conti pubblici non vengono riequilibrati. luogo, quest'anno, grazie a quella manovra, colpiamo anche un altro degli obiettivi, la cosiddetta crescita programmatica,

una connotazione di carattere recessivo. È evidente che in questo modo non si riuscirà

Questa è la grande preoccupazione che la lettura del DPEF, alla luce delle manovre concrete effettuate dal Governo, evidenzia. Non solo, ma è forte il silenzio di questo Documento sui temi che attanagliano

detto bene prima il senatore Sacconi: è evidente che la questione delle infrastrutture, e quindi del concentramento di risorse per tale obiettivo, non viene presa in adeguata considerazione. Così come non viene preso in adeguata considerazione il problema dell'energia. Sono delle strozzature grandi che vanno affrontate con scelte coraggiose delle quali il Governo non può farsi carico in ragione delle sue grandi contraddizioni interne. Si nota qui, dunque, il *deficit*, anche politico, di questo Governo. Non può prendere iniziative serie sull'energia, non può prendere iniziative serie sulle infrastrutture perché è attanagliato da gravi contraddizioni interne.

della competitività e dello sviluppo, ci propina la solita manovra: più tasse, più entrate (perché in questo modo si risanano i conti pubblici) e poi, forse, riprenderà lo sviluppo. Questa concezione ci pare del tutto inadeguata all'attuale situazione italiana.

la gente, nella gente, nelle istituzioni, nel Parlamento, la Casa delle libertà è riuscita a far correggere, in maniera assolutamente prima non prevista dal Governo, quel decreto che pur rimane grave, in particolare sui principi di contrazione della libertà dei cittadini e delle imprese. Sono state però fatte precipitose ritirate: penso alla questione dell'IVA sugli immobili, penso alla quantificazione della stessa e penso anche alla cosiddetta retroattività della possibilità di indagine.

*(Ulivo)*. Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, il Documento di programmazione economico‑finanziaria risulta significativo per le politiche di risanamento che pongono attenzione alle aree sottoutilizzate del Paese, ma un poco meno per efficaci azioni di indirizzo politico volte a sostenere il Mezzogiorno. I contenuti proposti dal DPEF al riguardo sono tali da prefigurare una futura evoluzione coerente con quanto affermato nel programma che l'Unione ha proposto ai cittadini, ma dovrebbero delineare le premesse per una strategia di interventi da attuare nei prossimi anni per il definitivo risanamento del Paese e per tentare di affrontare in maniera stabile la questione del Mezzogiorno. Il DPEF dovrebbe puntare a politiche di sviluppo del Sud Italia, con particolare riferimento all'impiego di misure utili a far ripartire il Mezzogiorno, alla riduzione del cuneo fiscale e alla programmazione di nuovi interventi infrastrutturali per colmare lo svantaggio competitivo, non solo con il resto del Paese, ma con gli altri Stati comunitari. Il contesto politico ed economico in cui questo Governo si trova costretto ad operare in merito alla situazione economica e finanziaria dell'Italia non è affatto tranquillizzante. Basti ricordare i dati contenuti nella relazione annuale SVIMEZ assai allarmanti, soprattutto riguardo la situazione nel Sud Italia. Il Mezzogiorno, infatti, dopo oltre dieci anni di crescita, lenta ma continua, sperimenta segnali di recessione. Stando infatti ai dati del 2005, a livello nazionale, secondo le stime dell'ISTAT, il PIL è rimasto fermo allo zero per cento, in calo rispetto allo scorso anno. A livello territoriale la forbice Nord-Sud si è allargata: il Centro-Nord conferma il dato nazionale di una crescita inchiodata allo zero per cento, mentre il Sud segna un meno 0,3 per cento. Si è così interrotta la fase, iniziata nella seconda metà degli anni Novanta, che ha visto il tasso di crescita del Mezzogiorno superiore a quello del Centro-Nord. È ormai di tutta evidenza come sia indispensabile effettuare, senza ulteriori ritardi, un' inversione di tendenza. Le positive reazioni di Bruxelles in merito ai contenuti del DPEF, anche alla luce dei provvedimenti di riforma delle professioni e dell'intervento strutturale di liberalizzazione in atto in Italia, pongono condizioni indispensabili per ottenere dalla Commissione europea l'assenso definitivo all'applicazione di quella fiscalità di compensazione che rappresenta uno strumento importante per la crescita e lo sviluppo del Sud e che dovrà essere posto come elemento cardine su cui incentrare le politiche fiscali per il prossimo quinquennio in favore delle aree sottoutilizzate del Paese e del Mezzogiorno in particolare. A tal proposito ritengo utile sottolineare come in merito al tema della riduzione del cuneo fiscale e contributivo gli interventi di riduzione dovrebbero essere prevalentemente destinati alle imprese che investono nel Mezzogiorno, proprio perché si tratta di interventi diretti a recuperare competitività di costo e quindi a favorire lo sviluppo. Condivido, infatti, le preoccupazioni di chi ha affermato che un'applicazione diversa di detta norma contributiva, determinerebbe un effetto assai sfavorevole per il Mezzogiorno; conti alla mano, i risparmi sarebbero del 67,5 per cento al Nord, del 23 per cento al Centro e solo del 9,4 per cento al Sud: un'operazione dal forte sapore antimeridionalista che tradirebbe le determinazioni di fondo cui si ispira la linea di Governo. La politica di sviluppo e coesione a favore del Mezzogiorno deve essere finalizzata ad accrescere la competitività dei territori regionali che presentano una sottoutilizzazione delle proprie risorse, non solo attraverso una sorta di compensazione dei divari di sviluppo, ma anche e specialmente finanziando le azioni che accrescono l'offerta di beni e servizi pubblici e migliorano le condizioni di contesto. In merito al tema del trasporti va sottolineato come si è creata una forte aspettativa per un rilancio della politica e della pianificazione di settore, le quali entrambe, negli ultimi anni, nonostante alcuni risultati positivi, hanno perso oggettivamente peso rispetto alle infrastrutture. Allo stesso tempo, è necessario mantenere uno stretto legame fra politica dei trasporti, della logistica e della programmazione infrastrutturale, affinché le decisioni di investimento in opere pubbliche assumano una concreta priorità e siano funzionali a un disegno strategico volto allo sviluppo logistico del Paese. Più in generale è importante rilanciare le misure a sostegno del combinato strada-rotaia e rotaia-mare ed una maggiore e più specifica attenzione deve essere dedicata agli interporti, la cui diffusione risulta deficitaria in tutto il Paese e, in particolare, nel Mezzogiorno. Anche in questo ambito devono prevalere le logiche di sistema e di integrazione logistica, favorendo la realizzazione di infrastrutture effettivamente necessarie e il loro collegamento in rete. Aggiungo un breve richiamo alla strategia che viene proposta nel DPEF per promuovere lo sviluppo del Mezzogiorno e delle altre aree sottoutilizzate. Il Documento evidenzia come risulta necessario sviluppare politiche volte ad incrementare gli investimenti piuttosto che gli incentivi all'investimento. Nello scenario programmatico delineato, però, la spesa in conto capitale del Paese rimane invariata, e sale la quota del Mezzogiorno, ma si segnala negativamente come l'obiettivo indicato per il periodo 2007-2011 di portare la spesa in conto capitale nel Mezzogiorno al 42,3 per cento del totale determini di fatto il sostanziale abbandono dell'obiettivo del 45

come sollecitazioni evidenziate per essere accolte. Non vogliamo una questione meridionale da contrapporre a una questione settentrionale, ma una questione nazionale che possa prevedere risposte differenziate.

presenta, per la verità con grave e colpevole ritardo da parte del Governo, un documento allegato previsto dalla legge n. 443 del 2001, la cosiddetta legge obiettivo, tanto contestata dall'attuale maggioranza parlamentare. Le ragioni di questa contestazione, che hanno accompagnato tutta la dialettica inerente l'ammodernamento infrastrutturale del Paese di questi anni anni (opposizione che si è accentuata in questi ultimi mesi di campagna elettorale), riguardano essenzialmente due aspetti. Il primo è che il valore complessivo del programma decennale delle infrastrutture strategiche fosse sproporzionato rispetto alle coperture finanziarie possibili. Su questo punto, stranamente, il documento presentato dal ministro Di Pietro compie una prima operazione verità: l'atto ricognitivo condotto dal Governo analizza in 58,471 miliardi di euro le risorse appostate disponibili, a fronte di 174 miliardi necessari per il complessivo piano decennale. Vorrei fare due semplici considerazioni: 58,4 miliardi sono circa un terzo del fabbisogno complessivo e questo fabbisogno è stato assicurato dal 2002 al 2006, cioè soltanto in quattro anni, quindi per circa 15 miliardi di euro l'anno. se questo Governo garantisse 15 miliardi di euro l'anno nei sette anni restanti per l'attuazione del piano decennale avremmo tutte le risorse disponibili. Da qui scaturisce scaturisce una conferma: che il piano predisposto dal precedente Governo fosse un piano realizzabile e subordinato soltanto alla volontà materiale di farlo. Il documento del ministro Di Pietro fa un'altra affermazione di grande rilevanza, sorprendente per quello che fino ad oggi aveva detto l'opposizione:

La seconda considerazione, di cui risente invece moltissimo l'allegato presentato, è che la frantumazione delle scelte ha disperso gli interventi in un quadro disorganico, quasi tramutandoli in interventi a pioggia. Basta invece a tale riguardo fare un'analisi molto semplice e guardare gli interventi attribuibili al corridoio 5, al corridoio 1, al corridoio Genova-Rotterdam, ai corridoi trasversali e ai nodi urbani (a detta di tutti priorità assolute nell'azione di ammodernamento del quadro infrastrutturale) per capire che il 95 per cento delle risorse è riconducibile a a questo tipo di pianificazione inserita in una più generale pianificazione europea alla quale il nostro Governo nel 2003 ha partecipato in modo determinante. Mi riferisco alle reti TEN e al piano europeo di ammodernamento delle infrastrutture di trasporto per consentire in modo fattuale la libera circolazione dei passeggeri e delle merci.

le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare». Dice poi che l'individuazione è operata a mezzo di un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (qui segnalo che manca

d'intesa con i Ministri competenti e le Regioni o Province autonome interessate; programma inserito, previo parere del CIPE - altro passaggio determinante - e previa intesa della Conferenza unificata, nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

scelti d'intesa con le Regioni e supportati da un piano su fonti e impieghi non limitato all'annualità ma alla triennalità. Ebbene, tutto ciò che obbligatoriamente per legge andava prodotto non è stato fatto. Proprio questa motivazione denuncia l'inutilità del Documento e al tempo stesso questa assenza programmatica, questo vuoto decisionale non consente nessuna valutazione su un'area strategica, quella legata all'infrastrutturazione organica del Paese che, se non elaborata in questa fase di esame e di approvazione del DPEF, rende monco in maniera sostanziale l'intero dibattito sul Documento di programmazione economico‑finanziaria.